Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale. Inoltre, il Governo ha espresso parere favorevole sulla mozione n. 93 (testo 2) dei senatori Tomassini ed altri, ha condizionato il parere favorevole sulla mozione n. 102, della senatrice Bianchi ed altri, ad una riformulazione ed ha espresso parere contrario sulla mozione n. 105, dei senatori Belisario ed altri.

siamo convinti di avere scritto una mozione che possa servire alla causa e siamo convinti che il Governo possa attingere qualche consiglio per poter operare al fine di debellare questa triste infezione.

in maniera chiara, perché comunque, sia quella a prima firma Tomassini, sia quella a prima firma Bianchi, pur essendo diverse dalla nostra, contengono delle richieste che noi approviamo.

programmazione questa infezione non la debelleremo), garantendo la riservatezza e il consenso informato, nonché la promozione di un ambiente sociale e giuridico favorevole. Ecco perché, signor Sottosegretario, ve lo chiede il Papa, ve lo chiedono i cardinali, ve lo chiede l'ordine dei medici, ve lo chiediamo anche noi, di modificare quella norma relativa ai clandestini,

un dogma, ma deve essere assolutamente favorito da uno Stato laico, pur nel rispetto di tutte le opinioni possibili e immaginabili presenti in questa Assemblea.

apprezzamento per la posizione assunta dal Gruppo che il senatore Astore rappresenta. Il Governo, ed in particolare la Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS, recepiranno, certo, gran parte dei contenuti della mozione Belisario. D'altra parte, però, il Governo non ritiene opportuno intervenire con iniziative volte ad espungere norme attualmente oggetto di esame parlamentare.

della entrata in scena di questa malattia, ad essere ancora qui, in un'Aula parlamentare, a presentare e votare una mozione che impegni il Governo a fare prevenzione. L'imbarazzo è dettato proprio dal fatto che così tanti anni sono passati e i dati che ci arrivano dalla Conferenza internazionale del 2008 sono tutt'altro che rassicuranti.

non si sottopongono al test e che in Italia la situazione sembra essere ancora più drammatica, non tanto nei valori numerici assoluti quanto percentualmente, se è vero che i sieropositivi sono stimati essere 130.000 e quelli accertati dai test 65.000, esattamente la metà. Questo è il punto su cui veramente bisogna riflettere ed il motivo fondamentale per cui credo si debba sostenere con forza, veramente tutti assieme, queste mozioni, anche se - ripeto - dovrebbero non essere nemmeno necessarie. Prendo atto delle parole del sottosegretario Fazio, pronunciate ieri in maniera molto positiva, di avere comunque riattivato la Commissione a livello ministeriale perché credo che sia veramente da lì che si debba ripartire per essere ancora più incisivi nella lotta contro l'AIDS. L'altro dato, su cui vorrei richiamare l'attenzione, è sull'evoluzione stessa di questa terrificante malattia che nei primi anni è andata a colpire sostanzialmente nicchie, emarginazioni della nostra società, fondamentalmente le tossicodipendenze, i tossicodipendenti. Dopodiché, questa malattia ha cominciato a diffondersi in tutti i settori della nostra società civile, omo ed eterosessuale, senza particolari suddivisioni. Poi vi è stata l'evoluzione in cui dal dramma della sieropositività si è passati alla speranza della terapia, della cura e non certo della guarigione, della possibilità di debellare questo virus, ma sicuramente della cronicizzazione della malattia e quindi ad una aspettativa di vita sicuramente più lunga, quasi normale rispetto agli individui non affetti da AIDS.

Soprattutto, credo sia fondamentale e vincente una corretta ed incisiva ulteriore campagna di informazione riguardo alla malattia e alle possibili conseguenze e, ancor più, alle possibilità di prevenzione. Il dato più drammatico

viene determinata in riduzione, pressoché in tutti i Paesi. Nel nostro Paese, invece, ci sono alcune situazioni, riportate in maniera emblematica quali quella del Lazio e della Toscana, dove l'incidenza della malattia tende ad aumentare. Credo che socialmente

qualora venga accettata da parte della collega Bianchi e degli altri firmatari la modifica proposta dal Governo, saremo prontissimi a votare anche la mozione presentata dai colleghi del Partito Democratico. anzi, l'occasione per esortare i colleghi ad accogliere questa modifica, perché sarebbe un peccato non condividere una mozione che contiene dei passaggi assolutamente unici, come quello della lotta all'AIDS dei minori e dei bambini, che credo sia veramente il futuro.

però presente un passaggio assolutamente inaccettabile per noi, lo stesso a cui faceva riferimento il collega Astore durante la propria dichiarazione di voto; su questo principio abbiamo delle visioni, ovviamente, diametralmente opposte.

un pronto soccorso. Mi spiace in parte che tale norma non sia stata da tutti compresa in tutta la sua sostanza; essa non vuole essere un qualcosa che va a limitare le possibilità di terapia e quindi la salute dei cittadini extracomunitari, anzi,

ad eventuale diffusione sociale che possono insinuarsi nella società, non solo dei clandestini ma anche dei regolari ed anche nella nostra.

diffusa perché non curiamo i clandestini, anzi fino ad oggi - e continueremo anche domani - essi vengono normalmente e direi sapientemente curati. Quando ho studiato medicina - e questo esame risale ormai ad una ventina di anni fa

individui extracomunitari e clandestini, che molto spesso vivono in condizioni perlomeno precarie, la tubercolosi se la portano appresso dai loro Paesi, un po' la diffusione di questa e di tante altri malattie favorita dalle condizioni igienico-sanitarie in cui versano e non certo dalle cure prestate dai medici nelle nostre strutture sanitarie. Ringrazio tutti ed esorto veramente l'Aula ad un voto unanime nei confronti di questa problematica sociale.

opportuno adottare misure finalizzate ad assicurare un'adeguata prevenzione, informazione e terapia nei confronti di tutti i cittadini stranieri.

Occorre fare dunque un esame realistico di quali siano anche i fattori culturali che favoriscono la diffusione di questa malattia: mi pare che ci sia una certa sottovalutazione del problema,

la nuova direzione della sezione HIV e AIDS della città di Washington ha promosso una campagna per favorire i test per individuare la diffusione di questa

tratta della stessa percentuale dell'Uganda e questo la dice lunga sul fatto che l'AIDS è anche un nostro problema.

e dobbiamo avere coscienza del fatto che la malattia non è stata né contenuta, né debellata. Andrebbe quindi forse fatta una riflessione a proposito dell'importanza della prevenzione. Sono passati 27 anni da quel 5 giugno del 1981, quando vennero per la prima volta resi noti i primi casi di AIDS. Vorrei ricordare che allora fu grazie ad una forte iniziativa delle associazioni omosessuali che si capì l'importanza della prevenzione per contenere la diffusione dell'infezione che a quel tempo non poteva essere curata e portava alla morte. Purtroppo questa azione è venuta progressivamente scemando e, nella stessa Conferenza del Messico del 2008, gli esperti hanno sottolineato come l'obiettivo prevenzione in questi anni sia diventato sempre più marginale rispetto all'obiettivo cura, mentre invece cura e prevenzione, essendo strettamente collegate, dovrebbero viaggiare insieme anche perché, a fronte di una riduzione dell'indice di mortalità, c'è un significativo aumento del tasso di sieropositività. Per ora altre possibilità non esistono: ci sono 25 vaccini in via di sperimentazione, tra cui uno anche nel nostro Paese, ma non si sa quali saranno i risultati che raccoglieremo da questa sperimentazione. Nel nostro Paese abbiamo messo in luce - come ricordato anche nella nostra mozione - il drammatico problema dei neonati e dei minori, e in questo abbiamo ripreso con forza una denuncia fatta dall'UNICEF. Occorre che le future madri vengano correttamente informate quali sono le modalità di trasmissione del virus; si favorisca presso queste giovani donne la diagnosi precoce, l'uso delle terapie che evitino l'aggravarsi della patologia e che ne impediscano anche la trasmissione ai nuovi nati. Nella risoluzione del Parlamento europeo del novembre scorso c'è un pressante invito agli Stati membri ad affrontare la prevenzione e l'informazione sull'AIDS, oltre che a migliorare le tecniche di sperimentazione e di trattamento della patologia. Il sottosegretario Fazio, nella risposta che ha dato ieri, ha sottolineato l'importanza della ricostituzione della Commissione nazionale per la lotta contro l'AIDS; lo ritengo un risultato positivo devo ricordare al Sottosegretario che ho visto il documento prodotto nel marzo 2008 dalla Commissione precedente che aggiornava le conoscenze sulle terapie dell'infezione dell'HIV. Penso sia importante a questo punto, anche sulla base delle mozioni che qui sono state discusse, che si faccia operare la Commissione per produrre un piano organico, Sottosegretario, come quello previsto dall'articolo 1 della legge 5 giugno 1990, n. 135. Sappiamo che quella legge per alcuni aspetti è superata, perché oggi

al Governo e alla Commissione per l'attuazione di un piano organico che riguardi prevenzione, informazione, ricerca, sorveglianza epidemiologica, sostegno all'attività del volontariato, attenzione alle nuove realtà della popolazione, agli immigrati, ai giovani, che sempre più precocemente entrano nella vita sessuale senza le corrette informazioni. Infine, vorrei chiedere anche al Sottosegretario che il piano generale della prevenzione, che è scaduto nel 2008,

Signora Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghe e colleghi, con la mozione n. 93 il Senato italiano intende rispondere alle richieste che le istituzioni europee hanno fatto agli Stati membri (in particolare con la risoluzione del Parlamento europeo del 21 novembre 2008 sull'HIV/AIDS: diagnosi precoce e cure tempestive, adottata all'unanimità) e vuole ribadire con maggiore forza l'impegno che chiede al Governo per affrontare un tema complesso e dalle delicate sfaccettature. La mozione che vi invito ad approvare non si limita a proporre considerazioni, a lanciare semplici dichiarazioni di principio, a ribadire triti auspici, ma vuole essere sprone ad azioni precise e puntuali nel modellare l'approccio europeo alla realtà della nostra situazione nazionale. Il primo passo concreto è la diagnosi precoce della sieropositività che si potrà ottenere solo attraverso la diffusione del test. La nostra convinzione si basa tra l'altro sulla valutazione in merito fatta dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, che lo scorso anno ha prodotto una relazione dal titolo «Il test HIV in *Europa***:** *dalle politiche all'efficacia», cui*, nel ribadire che l'HIV è una malattia trasmissibile con alti tassi di morbilità e mortalità, mette al primo posto tra le priorità per la prevenzione la spinta alla diffusione del test*,* con lo scopo di farlo diventare una parte normale degli standard di cura medica. Questa è un sfida strategica che ci sentiamo di condividere e che, se vinta, porterà anche a una fondamentale crescita culturale del Paese con la graduale eliminazione dello stigma sociale che ancora, purtroppo, aleggia sulla malattia. Sentiamo forte l'esigenza di tenere alta la guardia contro l'HIV/AIDS, che continua a mietere vittime in Italia come in Europa e nel mondo. Abbassare l'attenzione su un tema così importante per la salute pubblica ha, di fatto, generato una sorta di contagio inconsapevole provocato dalle persone infette non diagnosticate. L'accesso al test per l'HIV, e di elevata qualità, è essenziale, poiché nella maggior parte degli individui l'infezione da HIV rimane asintomatica. È una malattia seria che, non scoperta e non trattata, è trasmissibile sin dal primo giorno dell'infezione. Non è solo un problema di salute pubblica quello che vogliamo affrontare, ma anche di cura della persona malata ed ignara di esserlo. Stime del reparto di epidemiologia del dipartimento di malattie infettive dell'Istituto superiore di sanità dicono che in Italia esistono in realtà almeno 130.000 sieropositivi mentre i casi diagnosticati sono soltanto 65.000 esiste quasi il 50 per cento di sommerso). Il Centro europeo per il controllo delle malattie ribadisce che la consapevolezza della malattia attraverso la diagnosi precoce e l'accesso di *routine* ai test dell'HIV portano alla riduzione del numero delle diagnosi tardive; oltre alla diminuzione della diffusione dell'HIV, con la cura precoce si potrà tenere sotto controllo l'infezione nel paziente, tanto da non dare segni clinici evidenti e regalando al malato una vita normale e serena. Per questo motivo, la nostra mozione impegna il Governo ad agire per mettere in luce l'alto numero di persone che, senza saperlo, soffrono di HIV in Italia e alle quali è essenziale offrire la più ampia possibilità di effettuare il test, oltre che a promuovere la cultura della prevenzione per evitare che la malattia si diffonda. Vogliamo tracciare anche la via da seguire; nel nostro ordinamento esiste e lavora in maniera eccellente la Commissione nazionale per la lotta conto l'AIDS, organo tecnico del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, rinnovato nella sua composizione lo scorso gennaio e che vede, tra i propri membri, i massimi esperti in materia di HIV/AIDS del mondo scientifico e sociale. Richiediamo che sia proprio questa Commissione (ma il Sottosegretario ha già dato indicazioni positive in questo senso) in tempi ben precisi, ovvero sei mesi, a definire le linee guida nazionali per garantire, indurre e facilitare l'accesso al test. Non è un compito semplice, proprio per la sensibilità dell'argomento, che tocca aspetti, quali il diritto alla riservatezza, che devono essere sempre tenuti presenti e rispettati. Alla Commissione verrà affidato il compito di individuare i gruppi vulnerabili che dovranno avere una corsia preferenziale per accedere al test. questo un compito per il quale la Commissione è preparata a rispondere. Per ribadire l'impegno del Senato a riportare nell'agenda politica italiana il problema dell'HIV/AIDS, noi richiediamo anche di essere messi a parte del testo prodotto dalla Commissione. Questa mozione non vuole rimanere una bella lettura nell'albo d'oro del Senato e, proprio per questo motivo, impegniamo il Governo a monitorare l'applicazione di tali linee guida nazionali e a comunicarne lo stato dell'applicazione sul territorio nazionale attraverso una relazione annuale da presentare in Parlamento.

Il test e la cura precoci non solo prolungano ma migliorano la qualità della vita. Strategie innovative sull'accesso al test devono essere identificate, promosse ed applicate insieme all'attività di sostegno psicologico (pre e post test) quali parti integranti del processo di *testing*. Dobbiamo ricordare che l'HIV è un problema globale, europeo e italiano. Non perdiamo l'opportunità che sia proprio il nostro Paese a mettere in atto azioni concrete ed efficienti per la diffusione del test. sarà una testimonianza di eccellenza del sistema sanitario del nostro Paese da portare alla prossima Conferenza internazionale sull'AIDS, che si svolgerà a Vienna nel 2010. Voglio anche aggiungere che, pur apprezzando l'intervento del senatore Astore, riteniamo comunque di adeguarci all'espressione contraria del Governo per quanto riguarda

Prima di passare alle votazioni, avverto gli onorevoli colleghi che, in linea con una prassi consolidata, le mozioni saranno poste ai voti secondo l'ordine di presentazione e per le parti non precluse né assorbite da precedenti votazioni.

L'ordine del giorno reca: «Dibattito sugli strumenti della legislazione». Ricordo che, come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ciascun Gruppo ha a disposizione 20 minuti. Dichiaro aperto

La senatrice Finocchiaro ha posto in evidenza questioni che riguardano in generale il buon andamento dei lavori e la centralità del Parlamento come, ad esempio, la riduzione del numero dei parlamentari, l'utilizzo della decretazione d'urgenza, la modifica dei Regolamenti per il funzionamento di Senato e Camera e altro ancora.

come noto, si lega al problema della speditezza dei lavori parlamentari, con le note polemiche seguite alle dichiarazioni del Presidente del Consiglio voglio dire innanzi tutto che il Gruppo Lega Nord si compiace della maturata sensibilità di larga parte dell'opposizione. Invocare la riduzione delle poltrone comporta un'evoluzione politica che è nello spirito delle grandi riforme propugnate dal nostro movimento, anche a sanare l'annosa dicotomia tra Paese reale e Paese legale, riavvicinando le istituzioni ai cittadini. Solo per memoria, segnalo che il precedente Governo Prodi è stato quello con il più alto numero di Ministri e Sottosegretari nella storia della Repubblica. Duole peraltro ricordare che un drastico ridimensionamento dei parlamentari sarebbe stato diretta conseguenza di quella riforma della Costituzione varata dal precedente Governo Berlusconi

Considerato il precedente, non può che rallegrarci il progresso della sinistra nel comprendere ed accogliere alcune delle più diffuse istanze e necessità espresse dalla società civile, da quello che ho definito Paese reale, insomma dal popolo; è un processo politico che nell'opposizione appare anche serio e nondimeno faticoso e internamente contrastato. Per certi versi e su importanti temi vediamo una correzione di rotta e, a mio avviso, stona con questa ampia ed apprezzabile ricerca l'atteggiamento di fondo da monopolisti di verità monolitiche e indefettibili a cui la sinistra ci ha abituati per lungo tempo. Abbiamo ritrovato questa sconcertante attitudine negli anatemi scagliati contro il Presidente del Consiglio, accusato di pulsioni autoritarie, assenza di cultura costituzionale, incontenibile fastidio per le regole della democrazia, inossidabile visione proprietaria delle istituzioni, e via scomunicando. Più modestamente la Lega Nord ha semplicemente interpretato come una provocazione costruttiva e non come proposta fattibile l'idea di Silvio Berlusconi di limitare il voto ai soli Capigruppo, pur consentendo libertà di dissenso ai singoli parlamentari. La preoccupazione del *premier*,evidentemente, è una premura istituzionale che consiste nel desiderio di migliorare l'efficacia del Parlamento. Non è il *premier* ad avere creato il problema e neppure colui che lo ha sollevato per primo: avere evidenziato ildeficit di produttività parlamentare non dimostra disprezzo per la democrazia, semmai il contrario. Vogliamo estendere l'accusa di ducismo, ad esempio, agli autori di una ricerca comparata pubblicata da «Il Sole 24 Ore» nel luglio 2007 sulla velocità dei Parlamenti europei? Il Belpaese, oltre a possedere il record di parlamentari (952 contro i 905 francesi, i 638 tedeschi, i 609 spagnoli) vanta l'altro ben poco invidiabile primato, sempre a livello europeo, dell'improduttività legislativa. una situazione che richiederebbe dei correttivi di emergenza. Allo stesso modo, non deve stupire l'uso emergenziale della decretazione d'urgenza, strumento adottato proprio per uscire dal pantano delle lungaggini parlamentari. caso si punta il dito da un pulpito traballante, perché appaiono quanto meno zoppicanti le accuse di autoritarismo formulate formulate da chi, quando era maggioranza di governo, si guadagnò fama di avere espropriato il Parlamento con il ricorso sistematico alla questione di A quanti accusano questa maggioranza ed il Capo del Governo di attentare alla Costituzione ricordo che la decretazione d'urgenza è una prerogativa concessa all'Esecutivo precisamente dalla Carta costituzionale. Si tratta sicuramente di una corsia preferenziale, il cui accesso è regolato da un vigile eccellente cui compete la valutazione risolutiva sulla riconoscibilità degli elementi d'urgenza. Concludo ribadendo che qualsiasi proposta venga avanzata per migliorare l'efficienza del Parlamento in una prospettiva federale dello Stato deve essere ricondotta all'interno di un Parlamento sovrano che garantisca a tutto tondo la rappresentanza del territorio dello Stato e, soprattutto, democrazia e libertà, impedendo qualsiasi fuga in avanti da parte di chicchessia che metta in pericolo la democrazia compiuta di questo Paese. La Lega Nord sarà sempre vigile ed attenta affinché le libertà dei popoli vengano tutelate e salvaguardate.

sui rapporti fra il Parlamento ed il Governo e su questioni istituzionali di grande rilevanza fosse stato il presidente Schifani. Ce ne rammarichiamo e stigmatizziamo la sua assenza. La presidente Finocchiaro ha posto un tema serio, che riguarda non solo aspetti formali e costituzionali, ma che attiene alla vita democratica del nostro Paese. Sappiamo quanto abuso ci sia stato nella decretazione d'urgenza, nonostante l'articolo 77 della Costituzione

Maroni - che avrebbero meritato un coinvolgimento alle radici del Parlamento. Crediamo che questo modo di procedere non sia rispettoso del Parlamento e della sua centralità. Ma un aspetto che passa spesso in secondo piano è quello delle deleghe sotterranee, perché meno si nota. Da calcoli fatti, ci sono state circa 31 deleghe primarie su materie importanti: lavori usuranti, processo del lavoro, lavoro pubblico, sanità, Forze armate, industria e, da ultimo, il federalismo. L'articolo 76 della Costituzione lo consente, ma impone che il Parlamento vincoli il Governo all'interno di coordinate e indicazioni precise. Tutto ciò non è avvenuto e circa 20 di queste deleghe sono collegate alla finanziaria con indicazioni generiche, segno che la vera volontà è solo quella di spostare la competenza legislativa dal Parlamento al Governo. Deleghe addirittura introdotte di soppiatto, in Commissione o in Aula, con emendamenti. Pensiamo, ad esempio, alla delega sul processo amministrativo venuta fuori con un emendamento del Governo. Signora Presidente, le sembra questo rispettoso del Parlamento? nostro è un Parlamento relegato sempre a ratificare decisioni del Governo, giacché le iniziative parlamentari sono quasi inesistenti: qualche mozione o legge di cui il Governo non vuole assumersi la paternità. Eppure l'articolo 72 pone addirittura come soggetto proponente il singolo parlamentare sullo stesso piano del Governo. Per non parlare delle leggi *omnibus*, che mettono insieme argomenti diversi e che non consentono ai parlamentari di seguire, punto per punto, l'evoluzione legislativa. So quello che direte tra poco e quello che dirà, forse, il ministro Vito: anche voi avete operato nello stesso modo. Ci sono stati, signor Ministro, abusi anche in passato, anche se recenti sentenze della Corte costituzionale - la n. 171 del 2007 e la n. 128 del del 2008 - hanno ricordato con forza che dinanzi all'evidente mancanza di presupposti il decreto è da considerarsi nullo, anche se convertito dal Parlamento, che non può sanare un vizio che è all'origine. Ci sono stati i richiami del Presidente della Repubblica e del Presidente della Corte costituzionale, ma il problema è di natura politica, perché a differenza del passato è quello che il Presidente del Consiglio dichiara a gettare una luce negativa su questo modo di rapportarsi al Parlamento. Il presidente Fini ha fatto opposizione, anzi è stato uno dei capi dell'opposizione nei confronti del governo Prodi, ma non ha mai parlato di cesarismo, non si è mai preoccupato di richiamare il Governo al rispetto del Parlamento. E sappiamo che in ottobre lo stesso presidente Fini ha detto con chiarezza che se ci saranno abusi il Parlamento farà sentire la sua voce.

allora comprendiamo che il problema è politico e attiene ai fondamenti democratici del nostro Paese. Non lo dico per polemica. polemica. Vedete, questo Parlamento - è un'aggravante non di poco conto - non viene più eletto dal popolo, dai cittadini. Lo sappiamo bene e sappiamo anche che questa legge elettorale di fatto consente a poche persone di nominare il Parlamento. Se poi una di queste persone è il Capo del Governo, ciò costituisce una lacerazione fortissima e pone il Parlamento in una condizione di subordinazione nei confronti del Governo. Pertanto, non si possono considerare queste tessere del mosaico una ad una.

Ora, proprio perché non stiamo rivendicando nostre posizioni ma stiamo semplicemente cercando di fare rispettare fino in fondo le regole fondamentali che la Costituzione ci ha dato, la decretazione d'urgenza, dopo gli abusi che vi furono, dopo il fascismo è stata volutamente limitata dallo stesso articolo 77. Ebbene, dinanzi a tutto ciò, noi chiediamo alla Presidenza del Senato di assumere un'iniziativa forte come quella assunta dal presidente Fini perché il Parlamento sia rispettato, perché non sia considerato un orpello e perché si creda fortemente che il dialogo, l'interlocuzione, la collaborazione,

e per aiutare la politica del nostro tempo a rimanere fedele a quel patrimonio che i nostri padri ci hanno dato e che abbiamo il dovere politico e morale di trasmettere alle generazioni future.

credo che sarebbe riduttivo affrontare il tema solo ed esclusivamente con riferimento alla questione dell'abuso della decretazione d'urgenza e dell'espropriazione del Parlamento attraverso l'utilizzazione

l'attività di tutti i Governi che si sono succeduti nelle ultime legislature, in particolar modo da quando è cambiato il sistema elettorale nel 1994. È evidente che di un sistema istituzionale che è stato forzato ed adeguato al nuovo modo in cui si è organizzata la politica e il rapporto tra i cittadini e le istituzioni dal 1994 ai giorni

candidato. È quindi evidente che tutto ciò ha prodotto il risultato di caricare di aspettative superiori a ciò che istituzionalmente è consentito

a fare tutto ciò che vorrebbe in considerazione del fatto che il Parlamento ha i suoi tempi, che il Consiglio dei ministri ha i suoi tempi e così via. In proposito, signora Presidente, credo sarebbe opportuno

un Governo del Presidente - se così vogliamo definirlo - poiché la scelta dei Ministri è stata una scelta assolutamente discrezionale del Presidente del Consiglio, al di là

Di questi, 39 sono decreti-legge di cui 30 sono stati convertiti in legge,

ad intervenire con una possibilità d'iniziativa e di confronto successivi, cioè sulla scorta delle proposte che il Governo stesso ha avanzato. Analogo dato rileviamo con riferimento all'utilizzo del sistema delle leggi di delega: ci troviamo di fronte a 13 decreti legislativi

che anche il tema della questione di fiducia, che è stata posta dal Governo, se non ricordo male, per 13 volte (dieci alla Camera e tre al Senato), stia a dimostrare in buona sostanza che in quest'arco

di fatto, nella assoluta disponibilità del Governo, nel senso che esamina esclusivamente i suoi provvedimenti. Se così è, non vi possono essere alibi - è questa la considerazione di carattere politico - nel dire che i meccanismi regolamentari istituzionali sono tali da non consentire al Governo di portare a compimento il programma, perché vi è bisogno di un nuovo assetto istituzionale. Se tutta l'attività parlamentare, come dimostrano i dati, è assorbita è assorbita dall'attività e dalle proposte del Governo, significa che, avendo questo Governo una larga maggioranza, non può attribuire a nessun altro se non a sé stesso la responsabilità politica delle scelte e delle decisioni che assume e di quelle che non Questo è il primo dato che credo debba essere sottolineato e chiarito per evitare che si ricorra ogni volta a battute sul Capogruppo alla francese che vota per tutti, o sulla necessità di ridurre il numero dei parlamentari, salvo poi non farlo nella sede propria, cioè esaminando ed approvando una proposta di legge costituzionale che consenta di ridurre il numero dei parlamentari, considerato peraltro che c'è una larga maggioranza che consentirebbe di farlo senza andare al *referendum*, quindi con tempi rapidi e certi. [**Presidenza

Credo che su questo tema bisogna fare un'operazione verità e la verità è che dall'inizio della legislatura ad oggi il Governo, il Presidente del Consiglio e la maggioranza non hanno alibi, perché hanno tutti gli strumenti politici ed istituzionali per raggiungere, nei tempi

che sia opportuno, invece, fare una seconda riflessione, più di carattere istituzionale, che riguarda la circostanza che l'abuso della decretazione d'urgenza e l'espropriazione del Parlamento attraverso l'uso e l'abuso della delega è un fatto ricorrente, è un fatto che statisticamente interessa più Governi, bisogna dirlo con altrettanta franchezza ed onestà: nella passata legislatura, il legislatura, il ricorso alla decretazione d'urgenza non è stato minore, non è che il tentativo di utilizzare la delega legislativa per bypassare il confronto parlamentare non sia avvenuto riguarda anche le passate legislature, quando si sono alternati Governi di centrodestra e Governi di centrosinistra. Il problema è che è cambiato il modo - di questo dobbiamo cercare di discutere - di affrontare il rapporto fra l'Esecutivo e il Parlamento ed è evidente

che va sotto il nome di bozza Violante, che ebbe una condivisione, anche attraverso l'astensione dei Gruppi di opposizione del tempo, molto ampia. Da lì si potrebbe partire, per estrapolare alcune

introdurre una serie di correttivi che consentano di rendere più efficiente il sistema della decisione, così come dal 1994 ad oggi si è andato costruendo nel rapporto politico in questo Paese. L'altra questione riguarda la modifica dei Regolamenti parlamentari. Questo è l'altro tema che è oggetto di discussione e confronto anche nelle Giunte per il Regolamento ed è un tema che rischia di diventare una scorciatoia, se immaginiamo di introdurre surrettiziamente, attraverso un Regolamento parlamentare, le riforme istituzionali che non vogliamo

di voler modificare la Costituzione attraverso i Regolamenti parlamentari forzandoli oltre il limite consentito dalla Costituzione e ci concentrassimo, a Costituzione vigente, su quello che si può fare per migliorare il lavoro del Parlamento e del Governo, la prima cosa che dovremmo fare è

prevalente dell'attività del legislatore, riservando all'Assemblea l'assunzione piena della responsabilità politica sulle decisioni che riguardano i provvedimenti.

le votazioni sugli emendamenti, dovendo poi ricorrere, per velocizzare i tempi di esame di un provvedimento, all'*escamotage*di classificare quel provvedimento come collegato alla finanziaria e quindi applicare una tagliola e un regime di inammissibilità molto più stretto sull'esame degli emendamenti, per arrivare allo stesso risultato, cioè quello di di avere un provvedimento sostanzialmente definito in Commissione, che poi l'Assemblea deve votare non potendo che riproporsi solo ed esclusivamente gli emendamenti già presentati in Commissione. Usciamo allora dall'ipocrisia istituzionale e interveniamo sulle modifiche regolamentari partendo dal presupposto che l'attività legislativa luogo prevalentemente in Commissione e che l'Assemblea vota gli articoli e il disegno di legge finale, assumendosene la responsabilità. Questo è il senso, ad esempio, delle proposte di modifica delle proposte di modifica regolamentare avanzate dal mio Gruppo parlamentare. So ed ho letto che il Presidente del Consiglio - che non ha certamente accolto la nostra proposta - ha avanzato una proposta di questa natura e se non è l'ennesima battuta sui Capigruppo che votano per tutti, ma è una proposta seria, credo che da essa dovremmo partire. Peraltro, ciò consentirebbe anche di introdurre elementi di «moralità» della nostra attività ancora più ampi, perché invertirebbe anche il modo attraverso cui si lavora in questo Parlamento, obbligando obbligando i colleghi a fare ciò che dovrebbero fare cioè a stare tutti a lavorare nelle Commissioni di merito, ancorando anche - perché no, signor Ministro? - il pagamento di una quota della indennità

maggiore celerità nell'esame dei provvedimenti e un approfondimento reale degli stessi, effettuato in Commissione, e si metterebbe il Governo in condizione di non forzare, come spesso

senza dover fare ricorso alla decretazione d'urgenza. Un sistema siffatto, che si compone di poche modifiche regolamentari, consentirebbe di di essere in linea con la Costituzione e di fornire al Parlamento ed al Governo strumenti più efficaci e, al contempo, ai cittadini di avere un rapporto più trasparente anche con gli istituti parlamentari, evitando, ogni volta che vi è un elevato e sconsiderato numero di provvedimenti adottati dal Governo sotto i presupposti di necessità ed urgenza, di dover sempre e comunque intervenire per denunciare la forzatura istituzionale. Tutto questo, peraltro, porta anche ad un modo diverso di concepire il rapporto tra tra la politica e le istituzioni e consentirebbe in futuro di pensare ad un modo di organizzare anche la rappresentanza parlamentare, che non sia costretta nell'ambito di partiti che nominano i parlamentari. Più

più è semplice pensare che si deve tornare ad un sistema in cui l'elettore sceglie la propria classe dirigente, ad esempio, anche attraverso la preferenza, per cui ha un rapporto più civile, più corretto e più fidelizzato con le istituzioni. Lavoriamo, invece, sempre sugli annunci e continuiamo a forzare le norme costituzionali e regolamentari, fino ad arrivare in questa legislatura a configurare i decreti-legge, le leggi delega

fare lo slalom gigante tra il sistema delle inammissibilità di Camera e Senato per introdurre un emendamento che con un dato provvedimento non ha nulla a che vedere, ma che serve comunque a dare una risposta immediata ad un problema che emerge dal Paese. Dobbiamo cambiare questo sistema:

Il senatore Procacci con convinta passione ha richiamato tutti al rispetto delle istituzioni. Senonché ho sentito sentito nel suo intervento una contraddizione non modesta. Egli, infatti, nello stesso momento in cui si accingeva a parlare del rispetto delle istituzioni, si è rammaricato che ad ascoltarlo ci fosse soltanto un Vice Presidente del Senato, rappresentato dalla senatrice Rosy Mauro, in questo modo dando, a mio parere, segno di una certa volgarità nel rispetto delle istituzioni, perché qualsiasi Vice Presidente del Senato che segga in Aula è il Presidente del Senato.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Ministro, il Parlamento è l'organo rappresentativo del popolo per eccellenza, direttamente eletto dal corpo elettorale dunque, in quanto massimo organo rappresentante la sovranità popolare, viene prima di ogni altro organo statale per dignità politica. Si tratta di una preminenza di ordine politico che noi rivendichiamo e che vogliamo tutelare fino in fondo, combattendo l'antiparlamentarismo, purtroppo endemico, nella nostra società. La funzione costituzionale di rappresentanza generale della società, delle cittadine e dei cittadini, la funzione di rappresentanza politica del Parlamento, è per noi un dato irrinunciabile e rifiutiamo qualsiasi accusa, magari formulata dall'antipolitica qualunquistica, di un deficit di rappresentatività dell'attuale Parlamento, eletto invece con un sistema elettorale trasparente e che ha consentito finalmente di avere nella cosiddetta seconda Repubblica un sistema bipolare che funziona. Non siamo un corpo separato dalla società o, peggio, una casta, ma rappresentiamo con orgoglio la nostra comunità politica di elezione, cui rispondiamo quotidianamente e cui risponderemo alle prossime elezioni. Ciò che va corretto per noi è l'attuale assetto bicamerale del Parlamento, quel bicameralismo paritario nelle attribuzioni che mette in difficoltà anche il Governo che non è in grado di garantire la definizione di un'agenda coordinata dei lavori nelle due Camere; ciò incentiva l'uso frequente di strumenti non ordinari, quali il decreto-legge e la blindatura dei testi attraverso la questione dì fiducia. Noi vogliamo due Camere ma rappresentative di istanze diverse, un bicameralismo differenziato, con la creazione del Senato delle Autonomie. Questo nuovo bicameralismo federale, oltre a produrre benefici effetti in termini di rappresentanza delle istanze dei territori e dei popoli, produrrà anche l'effetto di velocizzare l'*iter* legislativo migliorando anche la qualità del prodotto finale. Da uno Stato interventista, anche sul piano legislativo, che vuole normare tutti i settori della vita umana occorre passare ad uno Stato federale leggero che, applicando il principio di sussidiarietà, faccia poche leggi chiare nei settori di competenza esclusiva statale. Che l'evoluzione storico-istituzionale abbia spostato il baricentro della forma di Governo parlamentare dal Parlamento ai Governo è ormai un dato di fatto riconosciuto non solo dai manuali di diritto parlamentare ma anche dalla classe politica. Il fenomeno dell'attività legislativa del Governo, nelle sue forme dell'attività delegata e della decretazione d'urgenza, va aumentando di pari passo con questa evoluzione storico-istituzionale. I decreti-legge tendono a divenire strumento ordinario di legislazione o, meglio, strumento privilegiato per lo svolgimento dell'indirizzo politico governativo. L'incremento, più volte denunciato in sede scientifica ed anche politica con toni scandalistici, dell'uso governativo della decretazione d'urgenza ci appare invece come l'esito di un processo evolutivo verso nuove forme di cooperazione tra il Governo e le Camere. Certo, il Governo non deve surrogare il Parlamento in quelle attività che sono specificamente dirette al controllo dell'Esecutivo o che comunque postulano l'alterità di Governo e Parlamento. Occorre allora trovare un bilanciamento tra la funzione costituzionale di rappresentanza del Parlamento e l'interesse del Governo - che, non dimentichiamolo mai, gode della fiducia del Parlamento - a governare attuando il programma in Parlamento. Se per raggiungere tale obiettivo occorra procedere ad una manutenzione dei Regolamenti, il nostro Gruppo è pronto a collaborare per scrivere queste nuove regole: un nuovo quadro di riferimento normativo regolamentare nel quale i movimenti e i partiti politici oggi presenti in Parlamento si riconoscano, indipendentemente dall'assunzione di ruoli di maggioranza e di Governo ovvero di opposizione. Proprio per tutelare il diritto del Governo a governare tra il 1988 e il 1991 è stato assegnato un ruolo prioritario al Governo nella decisione sulla programmazione dei lavori parlamentari. Evitiamo però che la pioggia dei decreti, di cui si chiede la conversione, impedisca una razionale programmazione dell'attività del Parlamento; ma questo è uno dei principali e più delicati compiti dei Presidente e del Consiglio di Presidenza, che ad oggi hanno saputo svolgere egregiamente con esiti felici. A nostro avviso, per dare maggiore efficienza alla macchina parlamentare, occorre valorizzare il lavoro nelle Commissioni permanenti, definite recentemente in un manuale di diritto parlamentare come i veri cavalli da soma del Parlamento. Elia parlò già nel 1961 del passaggio «dal Parlamento in Assemblea al Parlamento in Commissione», proprio per segnare la discontinuità tra i Parlamenti dell'Ottocento e quelli moderni. Forse, colleghi, 14 Commissioni permanenti sono davvero troppe e soprattutto occorre rivedere la ripartizione delle competenze, ferma al 1987. Dopo 22 anni è venuto il momento di riflettere sul numero delle Commissioni permanenti e sull'articolazione delle competenze, facendola aderire all'articolazione delle amministrazioni ministeriali. Le Commissioni permanenti sono i centri nevralgici dell'attività parlamentare e devono sempre più rappresentare l'interfaccia parlamentare dei Ministeri, evitando le degenerazioni del parlamentarismo. Chiudo con un accenno allo Statuto dell'opposizione, di cui spesso si sente parlare come la panacea di tutti i mali. A nostro avviso occorre indubbiamente dare valore al ruolo dell'opposizione, ma ciò richiede - e mi rivolgo ai colleghi dell'opposizione - anche uno sforzo culturale delle opposizioni. Le opposizioni, tutte le opposizioni, sino ad oggi hanno privilegiato la «cultura dell'emendamento», tendendo ad utilizzare ogni disegno di legge come occasione per introdurre nell'ordinamento norme ad esse gradite o per approntare imboscate parlamentari. La tattica emendativa forse davvero sta mostrando tutti i suoi limiti e comunque deresponsabilizza le opposizioni. Troviamo assieme, colleghi, nuove forme di collaborazione per valorizzare il ruolo dell'opposizione, rivitalizzando per esempio l'istituto della relazione di minoranza, incoraggiando le opposizioni a far emergere con chiarezza, nel confronto parlamentare, la propria posizione politica sul piano della proposta, con un atteggiamento costruttivo, superando la facile tattica emendativa e ostruzionistica, e magari costringendo anche la maggioranza a predisporre una relazione scritta, anziché affidarsi al meno impegnativo strumento della sola relazione orale. Siamo convinti che i tempi siano maturi per fare un passo avanti nella direzione di un Parlamento efficiente, la cui forza sia indissolubilmente legata alla forza del Governo e proceda di pari passo. Signor Presidente, colleghi senatori, signor Ministro, signori del Governo, un dibattito sui decreti-legge è in realtà, almeno in parte, un dibattito sulla debolezza del potere esecutivo nella storia delle istituzioni italiane: su quella condizione di sostanziale fragilità che accomuna il periodo statutario con la fase successiva al 1948, inaugurata con l'approvazione della Costituzione repubblicana. Nell'Italia liberale, infatti, nel momento in cui lo Statuto albertino venne a modificarsi grazie all'azione politica di Cavour e dei suoi successori, e dalla monarchia costituzionale si passò alla monarchia parlamentare, tra il re e il Parlamento, protagonisti rispettivamente della Costituzione formale e di quella materiale, il Governo si trovò ad occupare uno spazio residuale. Spazio che trovò proprio nell'arco di ponte che giungeva a descriversi tra queste due istituzioni, appoggiandosi, a seconda dei casi, ora più all'Assemblea, ora più al monarca, senza mai arrivare a coincidere del tutto con l'una o con l'altro. Da qui la necessità di Presidenze del Consiglio forti - Depretis, Crispi, Giolitti - e l'esigenza di quelle maggioranze variabili favorite dalla debolezza dei partiti, che nel lessico politico sono state degradate, un po' ingiustamente, a pratiche trasformistiche. Quando dopo la fine del fascismo si inaugurò il periodo repubblicano, ragioni storiche consigliarono di affievolire ulteriormente il ruolo e il potere del Governo. Per questo, pur rendendosi conto del difetto - andiamoci a rivedere gli atti della Costituente, in particolare della Seconda Sottocommissione - i nostri Padri costituenti evitarono qualsiasi legittimazione diretta dell'Esecutivo da parte della sovranità popolare. nella nuova temperie repubblicana, il Governo non poté neppure muoversi tra i due pilastri che ne avevano sorretto l'equilibrio durante la precedente stagione statutaria. Perché nel frattempo era venuto meno il re e, con esso, la sua fonte di legittimazione. Fu per questa ragione che il fulcro dell'architettura istituzionale venne assai presto a collocarsi al di fuori del circuito Governo-Parlamento, in quei partiti che almeno a partire dal 1953 ricoprirono di fatto la funzione di "stabilizzatori" del sistema politico italiano. Venuta meno la possibilità di muoversi lungo l'arco di ponte tra la Corona e l'Assemblea, i decreti-legge divennero così la valvola di sfogo dell'Esecutivo nei confronti dei partiti; rappresentarono, cioè, il vero punto di rottura rispetto all'ipotesi che giungesse a consolidarsi nel nostro Paese un vero e proprio regime di direttorio. Non è bastato a modificare del tutto questa situazione neppure l'evidente e ineluttabile declino che il ruolo dei partiti ha iniziato a subire già negli anni Ottanta e poi con la rivoluzione del 1994, la fine

i partiti hanno cercato di recuperare almeno una parte dell'antica forza nell'ambito della logica di coalizione. E questo ha indotto spesso le forze di maggioranza a concessioni di tipo "tattico" nei confronti di segmenti, soprattutto dei segmenti centrali dell'opposizione. Nonostante i profondi mutamenti, restava dunque attiva una pratica di concerto parlamentare che solo in parte si accordava con la logica e le esigenze del Governo. Anche in questo caso il decreto-legge è stato potremmo definirlo - un "bene rifugio" del quale l'Esecutivo ha potuto disporre per difendersi. L'esperienza del Governo Prodi, durante la quale la logica di coalizione è stata spinta fino all'esasperazione al punto di paralizzare addirittura il lavoro dell'Esecutivo, ha reso tutto questo drammaticamente chiaro. Oggi, dopo le elezioni dell'aprile 2008, ci troviamo a operare in uno scenario per certi versi nuovo e differente. La semplificazione del quadro politico, determinata dalle scelte autonome ma convergenti compiute a suo tempo da Berlusconi e Veltroni, ha portato il Governo e la maggioranza parlamentare, se non proprio a identificarsi, quantomeno a descrivere un *continuum*, soprattutto nel momento in cui ci si presenta di fronte alla pubblica opinione. E nel campo della controparte, seppure con ricorrenti tentazioni di delegittimare gli avversari e tornare a immaginarli come nemici, l'opposizione è stata spinta a presentarsi come Governo in attesa, interessata a contrapporre le sue proposte a quelle della maggioranza *pro tempore* e soprattutto a farle conoscere all'opinione pubblica. In tale contesto, signor Presidente, i decreti-legge sono divenuti lo strumento del Governo per realizzare il programma sul quale, insieme alla sua maggioranza, si è impegnato al cospetto degli elettori. Vi è dunque una motivazione nient'affatto secondaria che legittima il ricorso alla decretazione: quella di consentire alla volontà popolare di tramutarsi in azione di Governo. Nessuno mette in dubbio che si tratti di un mezzo improprio per raggiungere uno scopo non solo legittimo la soluzione non può consistere nell'ingranare la marcia indietro, gettando a mare tutto ciò che in termini di modernità politica il sistema ha guadagnato. Né si può immaginare di riattivare il vecchio concerto parlamentare al solo fine di recuperare margini di trattativa nei confronti del Governo. La storia dell'accumularsi del debito pubblico nel nostro Paese è fatta anche del ricorso a questa pratica. *(Applausi dal Gruppo* *PdL).* Se si vuole andare avanti, dunque, è necessario sottoscrivere un nuovo compromesso, un nobile patto tra Governo, maggioranza e opposizioni, perché la situazione attuale non giova a nessuno. In primo luogo non giova al Governo, che non può contare su una programmazione che garantisca efficienza alla sua azione. Mi consenta di dirle, signor Presidente, che non giova nemmeno alla maggioranza, che per conquistare camere di compensazione deve muoversi in sedi non istituzionali, e deve sempre guardarsi dal rischio che la sua funzione si riduca a quella di chi spinge il fatidico bottone. E non giova neppure all'opposizione, che da questo sistema non ricava nulla, se non l'effimera e in fondo mortificante soddisfazione di ritardare i lavori dell'Assemblea e far ricadere sul Parlamento, istituzione che sta nel cuore di tutti noi senza distinzione, il discredito che grava sulle istituzioni inefficienti, barocche, inadeguate a seguire il ritmo sostenuto imposto dai processi di modernizzazione. Da qui, signor Presidente, colleghi senatori, un appello a tutti i Gruppi presenti in questo Parlamento, nessuno escluso: scriviamo insieme un'altra storia, che possa dare prestigio all'istituzione che più di ogni altra ci sta a cuore, iniziando dalla riforma dei nostri regolamenti. Non vincoliamo la revisione delle regole di funzionamento delle Camere alla riforma della Parte II della Costituzione. Anzi: a maggior ragione se si intende lasciare che la modifica della Carta maturi in tempi adeguati, procediamo subito, insieme, ad un onesto compromesso regolamentare che risolva la crisi del processo legislativo, un'autentica emergenza a fronte delle problematiche con cui ogni giorno siamo chiamati a misurarci. Vi sono strumenti per assicurare al Governo tempi certi per la sua attività senza che tale razionalizzazione comprima lo spazio per l'approfondimento delle grandi riforme di sistema. Vi sono strumenti per garantire alla maggioranza la possibilità di esercitare una funzione critica anche nei confronti del suo Esecutivo, senza che questo assuma ogni volta i tratti della crisi di Governo. E vi sono strumenti per far sì che l'opposizione possa svolgere una più efficiente azione di controllo e garanzia, per restituire dignità alla sua insostituibile funzione istituzionale e rendere le sue proposte alternative più facilmente conoscibili dalla pubblica opinione. Su questi temi il Senato ha già attivato un confronto, e credo che da parte di tutti noi, maggioranza e opposizione, si debba gratitudine al presidente Schifani, che per primo ha mostrato sensibilità e sollecitudine. Tale pratica, però, non si può esaurire in una contrattazione privata tra i due maggiori Gruppi parlamentari. Di questo siamo assolutamente consapevoli. Così come stiamo compiendo ogni sforzo per autoregolarci e trovare una soluzione ai problemi di trasparenza senza che questo implichi uno stravolgimento delle nostre secolari prassi assembleari, allo stesso modo dobbiamo cercare in Senato di essere i primi nel concepire un sistema non roboante ma funzionale che riduca il *gap* di efficienza della nostra istituzione parlamentare avvicinandola ai cittadini e ai loro bisogni.

la discussione su questo tema presenta molteplici aspetti problematici. Cerco di tracciare un quadro minimo e sintetico dell'attività legislativa, ricordando

disegni di legge ordinari ma di iniziativa governativa, 19 sono disegni di legge di ratifica presentati dal Governo,

un parere non vincolante. Vi è una sola proposta di legge ordinaria rilevante, anch'essa di iniziativa governativa,

accantonando peraltro il cosiddetto decreto sicurezza da cui scaturiva in modo improprio, che è stato posteggiato su una corsia di emergenza. Si è verificata dunque la stranezza per cui una legge ordinaria è andata più veloce di un decreto-legge,

sulla lentezza parlamentare: quando il Presidente del Consiglio esige dalle Camere provvedimenti a suo vantaggio, il Parlamento è velocissimo e non si attarda Sarà attardato per altri motivi e sarà il caso di domandarsi per quali. Inoltre, l'attività parlamentare è incardinata essenzialmente sulla prevalenza, pressoché assoluta, dei decreti-legge.

Il decreto rappresenta una soluzione legittima, ma l'abuso della decretazione d'urgenza è stato stigmatizzato in due celebri sentenze della Corte costituzionale, concernenti la reiterazione dei decreti dei decreti e i requisiti di necessità e di urgenza. Siamo di fronte ad una prassi ormai entrata nell'uso, che ora forse è difficile smontare, ma che è contestata dalla disciplina.

una sorta di espansione impropria della portata normativa del provvedimento presentato, tanto che alla fine non si sa bene quali siano i suoi confini.

dimostra come il decreto venga sostanzialmente preso in considerazione e metabolizzato a scatola chiusa in Commissione e poi

del provvedimento di legge in corso, fino al punto da renderlo irriconoscibile. In tal modo, si determina un effetto negativo nei confronti della capacità emendativa dei parlamentari, i quali vedono trasformarsi il provvedimento sotto i loro occhi, qualche volta con emendamenti presentati in Aula in fotocopia, e

testi. In alcuni casi il Governo presenta solo in Aula emendamenti che modificano in modo pesante il testo in esame. Quale sarà la libertà di intendimento del parlamentare di fronte a questa metamorfosi processuale?

provvedimento una grave ed incongrua riforma della Corte dei conti. Questo giochino delle scatole cinesi, una dentro l'altra, è spesso ripercorso in altre occasioni e non va mai dimenticato, perché fa parte della tecnica

avvita all'interno dei provvedimenti legislativi le deleghe stabilisce alla fine un impaccio fondamentale. Decreti-legge da una parte e uso/abuso della delega dall'altra determinano una forma di trasferimento del potere legislativo dal Parlamento al Governo che si verifica prima e dopo: prima con la decretazione d'urgenza, dopo con la delega. All'interno di questa logica di trasferimento si devono tenere a mente i collegati *omnibus* che utilizzano la possibilità di richiamare materie eteroclite e congegnate all'interno di un provvedimento con cui hanno scarso rapporto.

dentro la legge e quindi compresso e probabilmente forzato anche nella logica. Si potrebbe dire che si passa dalla logica delle milleproroghe a quella delle milledeleghe. Significativo è il problema del codice ambientale e dei termini dei di riaprire i termini dei decreti correttivi del codice ambientale nonostante tali termini fossero scaduti da circa dodici ed il decorso di tale tempo determinasse la decadenza dall'esercizio della delega per espressa previsione della legge n. 308 del 2004, il Governo ha pensato bene di riattribuirsi una delega *ex novo*, senza principi e criteri ma facendo un semplice richiamo ai presupposti dai quali era decaduto per decorso del termine.

In questa maniera le Assemblee parlamentari vengono, di fatto, espropriate della funzione legislativa e talvolta capita addirittura che

Grazie, Presidente.

limitare il numero di ordini del giorno che ogni Gruppo può presentare ad un testo legislativo.

che va a toccare una delle ingombranti inefficienze del sistema, cioè il bicameralismo perfetto. Laddove potrebbe funzionare benissimo un monocameralismo specializzato per tematiche (materia che questa Assemblea ha già dibattuto

quella del federalismo sarà la vera fase dei cambiamenti radicali e sarà anche la vera fase di modernizzazione delle nostre istituzioni. Signor Presidente, ho ascoltato con attenzione l'intervento del senatore Quagliariello, come tutti gli altri interventi che lo hanno preceduto e seguito. Ho interesse a proseguire con il senatore Quagliariello l'analisi storica su come siamo arrivati all'attuale fase della produzione legislativa, ma lo farò in un'altra occasione.

viene da un'iniziativa proprio del Partito Democratico e debbo dire che osservando oggi il banco del Governo e osservando anche l'Aula, non propriamente piena, mi accorgo come

ritenendo inadeguati i meccanismi parlamentari ordinari, ha deciso di governare il Paese utilizzando quella decretazione d'urgenza che la Costituzione ha previsto come strumento eccezionale rispetto al monopolio parlamentare della legislazione. Precisamente questa è la questione che abbiamo sollevato e non è cosa di poco conto: stiamo discutendo se in Italia sia ancora in vigore la regola fondamentale di tutte le democrazie parlamentari, ovvero la separazione del potere legislativo da quello esecutivo. Sostenere che per approvare un disegno di legge il Parlamento non impiega meno di otto-nove mesi è

non sono numeri normali e se questo dibattito si fosse svolto tra qualche giorno, questi numeri sarebbero ancora maggiori. La decisione di governare con la decretazione d'urgenza, lo ha ricordato poco fa anche il senatore Quagliariello, è una decisione chiara, e ripetutamente esposta dallo stesso presidente Berlusconi. Cito: «Per risolvere la crisi abbiamo solo la decretazione d'urgenza». "È mia intenzione procedere con decreti-legge in ogni materia che riterrò necessaria". "Le difficoltà non si possono superare con i disegni di legge, ma con la decretazione d'urgenza". "Il *Premier* non può dare ordini, ma tutto si basa sulla sua autorevolezza personale, ha un solo strumento: il decreto-legge". "Il decreto-legge è l'unico metodo che abbiamo per governare". Sono tutte frasi del presidente Berlusconi e ricordarle può aiutarci ad avere piena consapevolezza che i 39 decreti non corrispondono a 39 casi isolati, a 39 emergenze improvvise, a 39 urgenze che il Governo ha dovuto regolamentare in tutta fretta. No. No. Siamo davanti ad una politica precisa, ad un metodo di governo impensabile soltanto sino a dieci mesi fa, che ha come obiettivo la distorsione dell'impianto costituzionale della formazione delle leggi. si tratta di una questione di smisurata importanza ed è grave che solo ora il Parlamento l'affronti direttamente ed esplicitamente. Vito, che il presidente Berlusconi non sia oggi qui in Senato. La ringrazio di essere qui, ma sono certo che anche lei comprenderà la nostra insoddisfazione profonda per l'assenza del Presidente del Consiglio. Senza il presidente Berlusconi questo dibattito perde gran parte del suo senso ed è infatti proprio il modo in cui il Presidente guida il Governo l'argomento di cui stiamo parlando e da lui personalmente dovremmo ascoltare delle risposte. Siedo nei banchi dell'opposizione, ma ho sempre rispetto per la figura del Presidente del Consiglio e quindi è rispettosamente che gli dico che sbaglia a snobbare così sfacciatamente il Parlamento. Sbaglia non solo per la considerazione che al Parlamento è sempre dovuta, ma anche perché comportandosi così non fa il suo personale interesse politico. Il confronto con l'opposizione può essere molto utile al Governo: ne migliora l'azione, ne aumenta il prestigio, ne accentua l'autorevolezza. Dirsi le cose in faccia è sempre meglio che nascondersi. Voglio sgombrare subito il campo da due argomenti che considero minori anche se sono rilevanti:

non intende modificare i Regolamenti parlamentari pur di non aiutare il Governo. Sulle lungaggini, Presidente, vorrei invitare il Governo e la sua maggioranza a guardare attentamente in casa propria. È significativo che il Governo emani decreti-legge così imperfetti e incompleti da indurre permanentemente maggioranza, relatore e Governo stesso ad emendarli dal momento in cui arrivano in Commissione, sino al momento in cui l'Assemblea li approva. dell'ultimo decreto, quello sullo sviluppo economico, abbiamo visto più di 350 emendamenti del Governo, della maggioranza e del relatore tra Commissione e Aula ed è così che i tempi si dilatano e la qualità delle leggi diventa infima.

interessa la presenza dei suoi parlamentari in Aula. Ed è significativo che Berlusconi abbia sostenuto la necessità di far votare i Capigruppo mentre parlava ai suoi deputati e senatori e ricordava loro che pochi giorni prima «63 parlamentari» «63 parlamentari» - suoi parlamentari - «invece di lavorare mi volevano mandare a casa e non si sono presentati all'ultimo voto di fiducia». Questo diceva Berlusconi colleghi, è possibile che, scava scava, forse alla fine emergerà che Berlusconi ha chiesto che voti solo il Capogruppo per normalizzare la sua maggioranza, non per sveltire il lavoro del Parlamento. Vi è poi il tema della revisione dei Regolamenti di Camera e Senato. L'abbiamo chiesta per primi. Nei fondamentali, la proposta di modifica sottoscritta dalla Presidenza del nostro Gruppo è uguale a quella che presentammo già nella XIV legislatura e che allora la Presidenza del Senato non sottopose mai all'attenzione della Giunta per il Regolamento. Ora il centrodestra ci chiede che il Regolamento garantisca al Governo e alla sua maggioranza gli strumenti necessari per realizzare il proprio indirizzo politico. Il Partito Democratico comprende questa richiesta ma ricorda che il suo consenso è rigidamente subordinato all'approvazione contestuale di nuove regole che assegnino all'opposizione adeguati spazi spazi di Aula, oggi, in questa legislatura nulli, e soprattutto efficaci strumenti per l'esercizio del diritto di controllo, oggi assolutamente inesistenti. È solo in questo quadro che potrà essere affrontato il tema dei tempi certi per i provvedimenti, cui il Governo, la maggioranza ed anche l'opposizione attribuiscono particolare urgenza. Ma mai, signor Presidente, potranno essere contingentati i tempi di discussione delle grandi leggi di sistema, delle riforme organiche, delle questioni di principio, delle leggi elettorali, delle leggi costituzionali. E aggiungo *ad abundantiam* - perché ne è già stato fatto cenno - che il Gruppo del Partito Democratico considera necessario che la riforma del Regolamento avvenga contemporaneamente alla riduzione del numero dei parlamentari ed alla revisione dei nostri Calendari di lavoro. Solo dando più tempo al lavoro delle Commissioni e diminuendo il numero dei senatori la riforma del Regolamento potrà dare buoni frutti. Ho apprezzato, signor presidente Schifani, l'auspicio che lei recentemente ha formulato e ripetuto più volte per una riforma del nostro Regolamento largamente condivisa. Suggerisco, però, di non mettere in relazione la riforma del Regolamento con il ricorso alla decretazione d'urgenza. Non sono i Regolamenti di Camera e Senato a costringere il Governo a produrre decreti su decreti. I decreti-legge sono legittimi solo se emanati nelle condizioni, assolutamente vincolanti, previste dall'articolo 77 della Costituzione. E considerare il decreto "l'unico strumento che abbiamo per governare", come dice il presidente Berlusconi, è incostituzionale. Non è, senatore Quagliarello, improprio, come lei ha sostenuto poco fa, ma incostituzionale! che attraversa una fase di profondo squilibrio istituzionale, sottende la presenza nel pensiero del Governo di una ben precisa concezione dell'organizzazione dello Stato, molto diversa da quella prevista dalla Costituzione. La domanda che dobbiamo porci, colleghi, non riguarda solo la legittimità costituzionale di ogni singolo decreto-legge, ma la legittimità della decretazione d'urgenza elevata a metodo di lavoro del Governo con il sovrappiù di un accavallarsi di maxiemendamenti, di emendamenti presentati all'ultimo minuto e quindi non esaminabili con la dovuta cura; di voti di fiducia richiesti non più solo per verificare la tenuta della maggioranza, ma per tagliare il dibattito parlamentare ed affrettare i tempi di approvazione. Più deleghe senza limiti e più il proliferare di leggi milleproroghe e di provvedimenti *omnibus*, dove entra tutto e il contrario di tutto! È questa, signor Presidente, l'ordinata strumentazione della legislazione voluta dalla nostra Costituzione? È questo un modo corretto per produrre leggi di qualità? Siamo certi che basterà qualche modifica ai Regolamenti parlamentari per far cessare questo andazzo? Credo sinceramente di no. I nuovi Regolamenti non basteranno almeno fino a che il sistema politico italiano non cambierà mentalità. In tutto il mondo sono in atto grandi cambiamenti. E alla fine della crisi anche l'Italia sarà molto diversa. Potremo uscire più forti o più deboli. Dipenderà da come sapremo affrontare la crisi e, soprattutto, se l'affronteremo in un clima di coesione nazionale e non cercando di ingannarci l'uno con l'altro. Se sapremo essere uniti, la crisi potrebbe essere una opportunità, una grande opportunità per cambiamenti positivi. Divisi affonderemo. Affonderà l'Italia. Il presidente Berlusconi sta sbagliando. Pensa che sia funzionale ai suoi interessi politici approfittare della crisi per modificare in profondità, da solo, contro metà del Paese gli assetti complessivi dell'ordinamento repubblicano, compresi i rapporti tra potere esecutivo e potere legislativo. La disinvoltura nell'uso dei decreti-legge è una parte di questo progetto. Il presidente Berlusconi sta cercando di cambiare la Costituzione senza modificarla, senza dirlo, con quotidiani aggiustamenti delle prassi e dell'interpretazione delle norme (si potrebbe dire che c'è un uso illegale del potere legale, una distorsione del significato della rappresentanza politica, con quotidiani sconfinamenti), assolutamente incurante delle contraddizioni. Ad ottobre il Presidente va a Napoli e dice che c'è sempre il Capo dello Stato che deve verificare se ci sono i requisiti di necessità e urgenza dei decreti‑legge; ma a marzo va a Cernobbio e cambia idea e, male interpretando la Costituzione, sostiene che la verifica dei requisiti di urgenza è sua responsabilità e il Capo dello Stato non può intervenire. Aveva ragione a Napoli ed aveva torto a Cernobbio. La debolezza e la contraddittorietà delle sue argomentazioni le rendono particolarmente irrispettose, ormai lo si percepisce chiaramente. si percepisce chiaramente. Il presidente Berlusconi ha in mente una profonda trasformazione del nostro Paese, delle sue istituzioni, della stessa società e della cultura nazionale e ritiene di disporre di mezzi sufficienti per attuare il suo disegno. È capo assoluto del Governo, con pieni poteri sui Ministri; dispone di un fortissima maggioranza parlamentare che lo garantisce totalmente. È proprietario o esercita grande influenza sul sistema dei *media*, a cominciare dalla televisione, come stanno a dimostrare i veti di questi giorni alla candidatura di eccellenti professionisti alla presidenza della RAI. Ha un consistente potere di condizionamento sull'economia, che esercita con assoluta discrezionalità, approfittando della crisi, anche su banche e grandi industrie. Laddove non riesce di comandare si adopera per dividere, come cerca di fare con il sindacato, o per neutralizzare, come cerca di fare con l'opposizione parlamentare. Il modello istituzionale cui sembra aspirare è di tipo presidenzial-plebiscitario, un modello che già occhieggiava nella riforma bocciata due anni fa dal*referendum* e che prevedeva addirittura lo scioglimento anticipato del Parlamento disobbediente. Ed hanno bluffato, mi dispiace doverlo dire, i senatori Gasparri e Bricolo, quando, giorni fa, hanno accusato in Aula il Partito Democratico di aver voluto il *referendum* del 2006 per impedire la riduzione del numero dei parlamentari: quel *referendum* fu voluto e vinto per altri motivi, fu voluto contro l'attacco del Governo e del centrodestra al principio della divisione dei poteri, contro la scomparsa di qualsiasi meccanismo di riequilibrio e garanzia.

il Presidente della Camera o il Governatore della Banca d'Italia, deve essere battuto e se possibile espulso dal sistema. Questo progetto il presidente Berlusconi non lo nasconde e lo proclama continuativamente la progressiva erosione attraverso l'uso della decretazione d'urgenza delle prerogative di quello che lui è arrivato a chiamare "super Parlamento" è solo uno dei pezzi del disegno. Ed è proprio a questo disegno che il Partito Democratico si oppone: lo consideriamo un pericolo grave per la democrazia italiana. È un disegno che (prendo ancora in prestito dal senatore Pera qualche parola) erode la natura democratica del nostro sistema. Il Partito Democratico - e ho terminato - fa opposizione usando gli strumenti che la democrazia parlamentare gli consente di usare. Non è un'esagerazione, né un assurdità aver chiesto al Presidente del Consiglio di partecipare personalmente ad un dibattito sulla questione centrale di ogni democrazia: il modo di fare le leggi. Considero un irrinunciabile diritto - e sottolineo diritto - dell'opposizione chiedere che il Capo del Governo venga in Aula per esporre ai senatori qual è la sua idea moderna di divisione dei poteri, qual è la sua concezione della democrazia. Che venga a smentire chi dai suoi comportamenti deduce una visione presidenzialista senza contrappesi, oligarchica e plebiscitaria, contrapposta a quella parlamentare. La mancata presenza del presidente Berlusconi in questo dibattito sottrae al Senato un suo preciso diritto, quello di ascoltare il Capo del Governo. Essa fa seguito ad una sua assenza pressoché assoluta dall'Aula del Senato. È venuto due volte soltanto e per lui erano due atti dovuti: una volta per presentare il suo Governo e l'altra per omaggio all'onorevole Bossi, quando si votava il federalismo fiscale. In altri tempi il Senato si sarebbe ribellato a questa forma palese e ostentata di disprezzo del Parlamento.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, il dibattito odierno assume una sua oggettiva rilevanza politica, benché non porti a decisioni operative.

per sottolineare ulteriori aspetti di natura politica, ai quali anche il senatore Zanda si è richiamato nella parte conclusiva del suo discorso. Innanzitutto vorrei dire al senatore Zanda, che ha citato una mia affermazione, che la confermo: sappiamo tutti che il*referendum* confermativo sulla riforma costituzionale, varata in Parlamento nel 2006 al termine di una legislatura importante, riguardava l'intero testo delle modifiche della Costituzione.

quell'occasione si è persa. Era legittimo non condividere quella riforma della Costituzione, che riguardava tanti punti; non contesto perciò il vostro diritto di aver espresso quella posizione nel *referendum,* ci mancherebbe!

perché approvammo quella riforma nella convinzione che entrasse in vigore, non per dire una cosa e farne un'altra. La mia affermazione resta dunque valida. Stiamo discutendo in realtà dei princìpi fondamentali di funzionamento della democrazia: questa è la realtà. Il Regolamento è importante, la riforma della Costituzione lo è ancora di più; ma il principio fondamentale che oggi sta soffrendo in Italia, e che forse soffre da tempo, è quello della democrazia, che vede la volontà popolare al centro dei processi di decisione.

senatore Zanda ha fatto riferimenti anche polemici alle affermazioni del presidente Berlusconi, il cui ossequio alla democrazia deriva dal fatto di rappresentare la maggioranza del popolo italiano, che lo ha scelto e lo ha votato più volte come capo di coalizione e di Governo, dato questo che non sfugge a nessuno:

Noi abbiamo un programma e lo stiamo attuando con la fatica e l'impegno che le regole parlamentari impongono, dall'economia alla giustizia, dai temi della sicurezza a tanti altri provvedimenti numerosi che sono stati già varati dal Parlamento. L'attuazione del programma è fondamentale affinché l'elettore, quando è chiamato nuovamente a votare, possa giudicare i Governi e le coalizioni in base a ciò che hanno fatto. Se però non è stato possibile realizzare il programma, non già per incapacità politica ma per la difficoltà delle regole, l'elettore giudicherà quella coalizione non per le sue colpe politiche ma per la difficoltà delle regole e allora il giudizio potrebbe essere negativo e impietoso. Noi riteniamo quindi ci sia la necessità di una revisione delle regole costituzionali e regolamentari nell'obiettivo di poter attuare dei programmi. alla polemica sui decreti, l'abbiamo fatta tutti a turno e non mi dilungo sulle cifre: voi ne citate alcune, noi ne potremmo citare altre (i voti di fiducia del Governo Prodi, per esempio); ma l'attuazione di un programma, anche attraverso un decreto o tramite un voto di fiducia, è la suprema espressione della democrazia e della volontà popolare quando è necessario tradurle in fatti e in norme. Potrei citare molti esempi, ma prendo un caso futuro di un provvedimento che ancora non è legge. Nel campo del piano casa e dell'edilizia la mia personalissima opinione è che un decreto dà maggiori certezze rispetto ad un disegno di legge. Quest'ultimo, infatti, viene discusso per un anno e nel frattempo i cittadini non sanno se i metri sono 20, 18, 15, quale tipologia

Vedete, quindi, come i concetti della necessità e dell'urgenza si modificano in una percezione condivisa. Noi riteniamo che si debba, nel rispetto delle regole fondamentali della democrazia, attuare la prima regola: consentire al popolo che vota di vedere attuato ciò per cui vota. Questa è la prima regola, quella che sta alla base di tutto: non c'è Costituzione, non c'è Regolamento, non c'è Parlamento e non esiste democrazia senza questa regola. Poi, che il Parlamento debba essere aggiornato e riformato non lo dico io qui, a conclusione di questo dibattito (poi interverrà il Governo ovviamente), ma lo dice un dibattito antico sulla Costituzione repubblicana. Circa il presidenzialismo, evocato prima con toni quasi sprezzanti, vi domando: oggi non c'è un presidenzialismo sostanziale? Secondo voi, gli elettori, trovando

che in pura teoria il Presidente della Repubblica, secondo la nostra Costituzione, potrebbe conferire l'incarico a chiunque altro; non avviene perché c'è una democrazia sostanziale che viene rispettata, ma noi non abbiamo ancora l'elezione del *Premier*, non dico una forma di presidenzialismo Credo allora che ci sia un ritardo nella riforma della Costituzione e dei Regolamenti rispetto a ciò che il Paese vive come una forma avanzata e moderna di democrazia decidente, che ha formato delle coalizioni, che vede nascere nuovi grandi partiti: è nato il Partito Democratico, sta nascendo il Popolo

riforma della Costituzione. A tale riguardo siamo aperti al dialogo e al confronto. È inutile fare una gara se sia meglio la bozza Violante o il testo da noi approvato nel 2006. I problemi sono la riforma del bicameralismo, il rafforzamento dei poteri dell'Esecutivo, la razionalizzazione dei lavori parlamentari per consentire alle minoranze spazi maggiori,

quale lei ha commentato alcune nostre proposte. Noi proponiamo, signor Presidente, che alcune proposte qualificanti del Governo possano essere portate in Aula con un termine temporale certo

quindi, un'invocazione al Presidente del Senato affinché la Giunta del Regolamento, non a caso presieduta dalla massima carica di questa Assemblea, possa intensificare il suo lavoro. Diamoci un calendario

senza vincolo di mandato, votando ciascuno per sé, ma soprattutto nel rispetto della volontà popolare e di quella democrazia che vede nel cittadino l'autentico principe e in noi gli strumenti di attuazione della volontà popolare, che è la prima regola ed espressione della democrazia.

Presidente, mi consenta di ringraziare lei, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi del Senato, ma anche il Gruppo del Partito Democratico, e il senatore Zanda

Questo è il tema al quale cercherò di attenermi, naturalmente senza sfuggire alle questioni, alle domande e alle critiche che sono state legittimamente sull'operato dell'Esecutivo, sulla scelta degli strumenti che il Governo ha inteso utilizzare in questo scorcio del primo anno di legislatura e sul rapporto che tale scelta ha avuto con l'attività del Parlamento.

e conseguentemente sono cambiate le aspettative e la percezione delle stesse che i cittadini hanno delle istituzioni, del Governo e del Parlamento. Non sono cambiate, però, le nostre regole e non sono conseguentemente cambiate le regole di funzionamento della democrazia, dell'attività parlamentare e dell'attività del Governo:

parlamentare, il Parlamento e le Camere avranno cercato di meglio corrispondere alle esigenze della nostra democrazia.

una limitazione ed una concentrazione esclusiva dell'attività e della funzione legislativa del Parlamento sul decreto-legge? Ciò ha determinato un'ulteriore compressione, quella della funzione legislativa propria ed esclusiva delle Camere?

in queste 41 sedute sono stati adottati 97 provvedimenti, dei quali solo 34, cioè circa un terzo, sono stati decreti-legge. Non c'è stato, quindi, un ricorso esclusivo o prevalente del Governo allo strumento del decreto-legge nell'ambito della propria attività legislativa. Ancora maggiore, naturalmente, è l'attività di altro rango e di altro genere del Governo; su questa però non mi soffermerò, perché non è stata richiamata dal dibattito. pertanto, di 34 decreti-legge: onorevole Zanda, lei ci potrà criticare per il numero dei decreti-legge adottati dal Governo Berlusconi, ma non certo per quelli adottati dal Governo Prodi che hanno impegnato l'attività del Parlamento in questa legislatura, perché credo che il numero citato comprendesse anche i cinque decreti adottati dal Governo Prodi nella fase conclusiva della sua attività. Vorrei fare un confronto con i precedenti Governi, soprattutto

anche questo aspetto - di non utilizzare tutti gli strumenti legislativi a sua disposizione ed anzi addirittura, onorevoli senatori, con una circolare dell'11 aprile 2007 (che non mi pare, senatore Zanda, abbia provocato scandalo, reazioni o occasioni di dibattito come quella in Parlamento), il presidente del Consiglio Prodi disse ai suoi Ministri di non ricorrere agli ordinari strumenti legislativi, ma di ricorrere solo ad atti amministrativi per evitare il confronto

dell'attività del Governo Berlusconi per rispondere ad alcune emergenze ereditate dal passato e assumiamo come periodo di confronto omogeneo, anche con lo stesso Governo Prodi,

l'idea che il Governo Prodi abbia costantemente varato meno decreti-legge rispetto al Governo Berlusconi viene ad essere smentita dalla realtà: in quel trimestre di avvio dell'anno 2007, infatti, il Governo Prodi varò ben sette decreti-legge; in questo trimestre il Governo Berlusconi ne ha varati solo quattro; e anche se consideriamo un possibile ulteriore decreto-legge in questa fase conclusiva del mese di marzo, siamo comunque al di sotto del numero di decreti che adottò il Governo Prodi. Grazie, che io mi sento non solo di non condividere ma anche di non poter né considerare né ammettere), sono stati rigorosamente vagliati nel rispetto dell'articolo 77 della nostra Costituzione e sono dotati dei requisiti di necessità ed urgenza,

ed improrogabili derivanti da situazioni giuridiche o legislative di fatto che si sono determinate, ed è questa una situazione rispetto alla quale tutti i precedenti Governi hanno dovuto corrispondere con l'adozione di decreti-legge, ad esempio quelli di proroga

Anche qui vengono in nostro soccorso alcuni dati. Le leggi approvate nella XVI legislatura dal sedicesimo Parlamento repubblicano in questi primi mesi sono state - come pure è stato ricordato - 58; di queste, solo 25 sono riconducibili a decreti-legge adottati dal Governo Berlusconi, cioè meno della metà. Quindi, i decreti-legge non hanno occupato in via esclusiva l'attività legislativa del Parlamento. E se è vero che le altre leggi derivano, comunque, da proposte del Governo, bisogna anche dire che questo corrisponde ad un'esigenza ormai diffusa in tutte le democrazie occidentali per le quali è l'iniziativa propria di proposta del Governo ad esaltare la centralità legislativa del Parlamento, per la ragione ricordata in diversi interventi: è solo attraverso la funzione di proposta legislativa che il Governo può cercare di attuare quel programma scelto dagli elettori e che è alla base del bene primario per il funzionamento delle nostre istituzioni, cioè la democrazia.

Ebbene, tre furono anche quelle giunte a compimento nella legislatura precedente, a dimostrazione di come ormai sia un dato consolidato degli ultimi decenni che il Parlamento si concentri su proposte governative. Ma l'esame di questi 34 decreti-legge, senza voler nulla togliere all'intervento del senatore Mazzatorta che ha parlato di un eccesso di cultura emendativa da parte del

proposti dal Governo Berlusconi all'esame del Parlamento sono stati modificati dal Parlamento stesso. Nessun decreto è stato approvato nella versione definitiva nello stesso testo con il quale era stato varato dal Consiglio dei ministri. Il potere di conversione e quindi il ripristino dell'attività legislativa propria del Parlamento è sempre stato esercitato coerentemente e correttamente da entrambe le Camere. Ai decreti-legge convertiti dai due rami del Parlamento sono state apportate circa 700 modifiche, la maggior parte delle quali proprio in questo ramo del Parlamento, al Senato. E l'origine di queste 700 modifiche è ampiamente e prevalentemente parlamentare, giacché solo 103 sono d'iniziativa governativa e quasi 600, invece, d'iniziativa parlamentare, come è giusto e corretto che sia. E di queste 600, oltre 100 sono addirittura di provenienza dei Gruppi parlamentari di opposizione. Quindi è stato esaltato il ruolo del Parlamento ed è stata ripristinata la sua funzione legislativa anche quando il Governo si è trovato nella condizione straordinaria di necessità e di urgenza di dover adottare atti che avevano immediatamente valore

Il Governo è stato messo nelle condizioni di dover ricorrere limitatamente a questo strumento straordinario in questo ramo del Parlamento. I colleghi di maggioranza e di opposizione, che a ruoli invertiti hanno vissuto l'esperienza delle precedenti legislature e di questa legislatura, sanno di cosa sto parlando. Nello stesso periodo dei primi dieci mesi di legislatura, il Governo Prodi al Senato della Repubblica pose sette volte la questione di fiducia; il governo Berlusconi l'ha fatto solo tre volte. Credo, quindi, che questo sia testimonianza di un diverso rapporto e rispetto del lavoro di questo ramo del Parlamento e delle Camere. Va aggiunto che complessivamente il numero di volte in cui è stata sinora posta la fiducia dal Governo Berlusconi, tredici, è perfettamente identico al numero

di esame dei decreti-legge per la quale non c'è un testo presentato dalla Commissione e il Governo deve comunque presentare un emendamento. Anche in questo caso (e non temo di essere smentito dai fatti e dagli onorevoli senatori), quando il Governo è ricorso all'uso estremo della presentazione di maxiemendamenti sui quali ha posto la fiducia, in quei tre limitati casi, l'ha sempre fatto nel rigoroso rispetto del lavoro parlamentare, in particolare di quello delle Commissioni di merito. Mi auguro in questo modo di aver smentito alcuni luoghi comuni sul presunto abuso del ricorso alla decretazione d'urgenza e sull'eventuale limitazione della funzione legislativa delle Camere.

i cui tempi sono noti a tutti. Mi permetto di aggiungere un altro dato, dal punto di vista del Governo. Sono ormai diverse legislature che si è consolidata l'accettazione di un dato di fatto, di una realtà che si ritiene essere insufficiente non solo per il Governo ma per lo stesso Parlamento, dire che giunge al voto finale delle Camere solo una minoranza dei provvedimenti che il Governo presenta all'attenzione del Parlamento.

questi temi, si pone quello dei tempi della decisione, che non è per spirito di fretta legislativa che il Governo pone, ma per uno spirito di adeguamento ai tempi della competizione internazionale. I tempi con i quali si assume una decisione, oggi fanno già parte dell'efficacia o dell'inefficacia della decisione stessa, per la velocità con la quale le decisioni vengono assunte e corrisposte e per l'esigenza che la società, la famiglia e le imprese hanno di avere risposte in tempi reali e conseguenti alla

modifiche regolamentari e costituzionali che il Parlamento intenderà promuovere e alle quali il Governo guarda con grande attenzione e fiducia. Sono stati posti alcuni temi dal presidente D'Alia e da altri autorevoli senatori sul ruolo e l'attività delle Commissioni, che giustamente devono essere esaltati nell'ambito delle prerogative costituzionali, nel rispetto del ruolo e delle funzioni delle opposizioni. Mi permetto di aggiungere anche che la centralità del Parlamento si esalta - fa bene

presentate sia dalla maggioranza che dall'opposizione. Bisogna uscire dal luogo comune che la centralità del Parlamento si realizza solo attraverso l'approvazione o no di emendamenti e di atti legislativi: si realizza anche attraverso la presentazione di atti di sindacato ispettivo e la votazione di indirizzi politici che il Governo - è stato corretto il richiamo del senatore Divina al rispetto degli ordini del giorno - è tenuto a rispettare. Questi problemi e non altri, senatore Zanda, ha inteso porre il presidente Berlusconi,

dalla Commissione bicamerale presieduta dall'onorevole D'Alema. Sono problemi all'attenzione del Parlamento da diversi anni, che con l'occasione di questo dibattito possono probabilmente trovare la spinta

Il Governo naturalmente da questo compito attende con fiducia la possibilità di meglio corrispondere alle esigenze dei nostri cittadini

perché le parole usate dal senatore Longo sono state disdicevoli e inappropriate, in primo luogo perché è mio costume sempre rispettare la Presidenza e i colleghi, ma soprattutto perché non tengono in alcun conto un aspetto: il Presidente del Senato non è soltanto colui che presiede l'Assemblea, è anche la seconda carica dello Stato. Mentre i Vice Presidenti possono sostituirlo nel primo compito, quello di presiedere l'Assemblea, è altrettanto vero che non possono sostituirlo nel suo ruolo di Vice Vice Presidente della Repubblica; tant'è vero che, in caso di impedimento del Presidente del Senato, è il Presidente della Camera, la terza carica dello Stato, che ne assume i poteri. Questa, caro collega Longo, era la ragione per cui chiedevo che il presidente Schifani fosse qui a presiedere la seduta si confrontava su un argomento di così grande rilevanza politica e istituzionale. Tant'è che la sua presenza, sia pur con un lieve ritardo, è stata poi assicurata all'Aula. Vede, Presidente, essere maggioranza non significa essere i padroni del Paese: significa esercitare un ruolo rilevante, quello di governo, in un equilibrio dei poteri garantito dalla Costituzione. a lei, signor Presidente, sento la rilevanza del fatto che lei è la seconda carica dello Stato. Non è una cosa in più. Lei non vota, il Presidente del Senato non ha mai votato per prassi, ma soprattutto perché, lungi dall'essere una figura di parte, è la figura che deve garantire la Costituzione e i Regolamenti. Perciò era importante la sua presenza e perciò faccio appello, dopo il dibattito che abbiamo svolto oggi, affinché, come garante delle istituzioni, ci faccia sentire in buone mani. Grazie, Presidente.

Grazie,

Quagliariello e Zanda quali sono i punti di contatto e qual è il lavoro svolto nelle ultime settimane, perché penso che la velocizzazione dei lavori parlamentari possa accompagnarsi

Detto questo, sono dell'idea che la velocizzazione dei lavori parlamentari passi non soltanto dalla modifica dei Regolamenti, ma dalla semplificazione del sistema istituzionale e parlamentare. Il bicameralismo sconta un prezzo, quello della duplicazione della lettura. È nato in un'epoca storica che ormai forse è cambiata e in ciò mi rifaccio ad alcune ad alcune osservazioni del presidente Gasparri, quando ha fatto riferimento ad una democrazia reale, diversa rispetto a quella formale scritta in alcune parti della nostra Carta costituzionale, che rimane comunque, ad oggi, il nostro faro e il nostro punto di riferimento. Con un'auspicabile riforma l'intento di tutti dovrebbe essere quello di creare una totale sovrapponibilità tra la Costituzione reale ed una nuova Costituzione formale.

Onorevoli colleghi, il 14 marzo di un anno fa, nella sua casa di Rocca di Papa, si spegneva Chiara Lubich, fondatrice e presidente dell'Opera di Maria, movimento ecclesiale conosciuto in tutto il mondo come il Movimento dei Focolari. Nata nel 1920 a Trento con il nome di Silvia Lubich, assunse quello di Chiara, sull'esempio di tante figure della tradizione cristiana, al momento della sua consacrazione con voti privati, avvenuta il 7 dicembre 1943. Determinante, per la sua radicale scelta di fede, l'esperienza degli orrori della guerra: poco più che ventenne, scelse di non rimanere con la famiglia, sfollata in montagna, ma di ritornare a Trento, devastata dai bombardamenti, e condividere la paura e la disperazione dei concittadini. In questo doloroso contesto, denso di fede e di coraggio umano, Chiara Lubich costituì, insieme ad un gruppo di amiche, il primo nucleo del Movimento, ispirato da una spiritualità incentrata sul tenace desiderio di incarnare nella società contemporanea la chiamata a tutti gli uomini ad «essere una cosa sola». Nasceva così il primo Focolare, espressione nascente di quella «spiritualità dell'unità» che nei decenni successivi Chiara Lubich avrebbe approfondito e meditato al punto da formulare proposte concrete, volte a permeare di questo spirito unitario tutti gli ambiti della società umana. Un momento fondamentale di questa evoluzione fu l'incontro, avvenuto nel 1948 a Montecitorio, tra Chiara Lubich ed Igino Giordani, luminosa figura di intellettuale e uomo politico, deputato della Democrazia Cristiana all'Assemblea costituente e nella prima legislatura repubblicana. L'adesione di Giordani al Movimento, oltre che sancire definitivamente l'apertura dei Focolari al contributo delle persone sposate, accentuò ulteriormente il carattere politico - nel senso più nobile della parola - della presenza ecclesiale e sociale espressa dai Focolari. Da questo fermento è nato, negli anni più recenti, il Movimento politico per l'unità, impegnato a diffondere la cultura dell'unità tra gli uomini e le donne che dedicano la loro esistenza all'impegno politico, senza limiti di appartenenza o di schieramento. Cuore della proposta è la riscoperta della fraternità come categoria politica, da porre sullo stesso piano dell'eguaglianza e della libertà, nel tentativo di ricomporre, in chiave cristiana, quel trinomio di valori posto alla base, sin dalla fine del XVIII secolo, di ogni moderno sviluppo della democrazia e dei diritti della persona umana. Tra i momenti di formazione, riflessione e incontro fra le diverse culture politiche proposti dal Movimento, meritano un particolare plauso e considerazione i percorsi di formazione politica rivolti alle giovani generazioni. Penso, in particolare, alle scuole di formazione alla cittadinanza avviate il mese scorso, ad opera del Movimento, proprio nella mia Regione, nelle città di Palermo e Catania. Il Movimento dei Focolari conta, oggi, più di 140.000 membri, ed oltre due milioni fra aderenti e simpatizzanti. È presente stabilmente in 89 Paesi del mondo e diffuso in altri 100. Ciò che più caratterizza il lascito di Chiara Lubich, rispetto ad altre realtà religiose ed ecclesiali, è la sua apertura alla partecipazione di persone provenienti da altre confessioni cristiane e addirittura da altre appartenenze religiose, come dimostra, ad esempio, l'appartenenza o la vicinanza al movimento da parte di migliaia di individui di fede islamica o buddista. Chiara Lubich, del resto, ha sempre affermato come il dialogo e l'unità abbiano sempre costituito la vera cifra dell'azione e dello spirito del suo Movimento, rivolgendosi, in particolare, in quattro direzioni: all'interno della Chiesa cattolica, nel dialogo ecumenico tra le diverse confessioni cristiane, con i seguaci di altre religioni, ed infine, con eguale convinzione ed efficacia, nei confronti di tutte le «persone di buona volontà» che esprimono convinzioni non religiose. La sua serena mitezza, che non si stancava di diffondere con un messaggio di pace e di unità, non è mai stata disgiunta dalle doti di tenace sensibilità e coraggiosa accoglienza, tipicamente femminili, che hanno sempre caratterizzato la guida e l'azione del Movimento, sin dalle sue origini trentine. Questo prezioso carisma è destinato a perpetuarsi nel tempo, per effetto degli Statuti dell'Opera, che prevedono che il Movimento continui ad essere presieduto da una donna, anche dopo la scomparsa della sua fondatrice. Nel ricordare Chiara Lubich, ad un anno dalla sua scomparsa, è allora doveroso rivolgere un caldo augurio di buon lavoro all'avvocato Maria Emmaus Voce, per molti anni tra le sue più strette collaboratrici, ed oggi presidente mondiale del Movimento, nell'auspicio che la memoria dei risultati - davvero straordinari -conseguiti in questi anni sul cammino della pace e dell'unità tra i popoli e le religioni, possa continuare a tradursi, come sta già avvenendo, in un rinnovato messaggio di speranza rivolto al mondo intero.

una delle persone che maggiormente hanno contribuito a gettare le basi per il dialogo interreligioso nel mondo. Da giovanissima, lo ha ricordato il signor Presidente, in estrema povertà, Chiara Lubich trova la sua vocazione in uno dei momenti più drammatici per la sua città: in una cantina, per scampare al bombardamento di Trento, con in mano solo il Vangelo e gli edifici che crollavano accanto a lei, capì, come ha amato ripetere più di una volta, che «ogni cosa materiale può crollare, ma non Dio, inteso come Amore». È proprio in quella occasione di difficoltà che si formò il cuore pulsante del futuro Movimento dei Focolari, che dapprima si dedicò all'assistenza dei malati e dei feriti di guerra e che poi percorse la strada spirituale del dialogo, arricchendosi di personalità come Igino Giordani, deputato democristiano che divenne cofondatore del Movimento, e del giovane Pasquale Foresi, il primo focolarino ordinato sacerdote. Fraternità universale, unità tra i cristiani, dialogo con le comunità ecclesiastiche non cattoliche, ricerca del confronto con altre religioni ma anche con i non credenti: erano questi i grandi obiettivi di Chiara Lubich e dei Focolari, che iniziarono col tempo ad avere una forte componente giovanile con il Movimento Generazione Nuova. Si riunivano in cittadelle di testimonianza, come quella di Loppiano, fondata nel 1964, mentre sempre più numerosi volontari si impegnavano nelle diverse realtà della società. Chiara Lubich si spese in prima persona per ricongiungere le confessioni di tutto il mondo in una grande famiglia: andò in Germania negli anni Sessanta e incontrò tutti i *leader* delle Chiese cristiane in un momento di delicati equilibri nei rapporti tra le confessioni. Parlò a Tokyo, davanti a diecimila buddisti, e a New York, davanti a 3.000 musulmani neri nella Moschea Malcolm X di Harlem, e poi presso la comunità ebraica di Buenos Aires, e ancora in India, per aprire il dialogo del suo movimento anche con il mondo indù. La sua apertura verso l'altro era sconfinata, non conosceva barriere né tabù. Soffriva, Chiara Lubich, delle grandi ingiustizie del mondo, delle disparità economiche tra le persone. Diceva, ancora una volta anticipando tutti nei tempi e nei temi, che "il terrorismo è frutto dello squilibrio tra ricchi e poveri", ma che «i beni non si muovono se non si muovono i cuori». Frasi che Chiara Lubich non lasciò isolate, ma che seppe concretizzare con proposte reali per cambiare il sistema economico consumistico di cui oggi tutti noi vediamo i drammatici effetti. Nel 1991 in Brasile, di fronte alla disastrosa realtà delle *favelas* lanciò la cosiddetta economia di comunione, trovando l'appoggio di centinaia di aziende che, come lei, condividevano l'idea di una diversa redistribuzione degli utili, che potesse interessare anche i più poveri, gli ultimi di ogni parte del mondo. Alla cultura dell'avere - diceva - bisognava sostituire la cultura del dare. Le sue iniziative trovarono l'attenzione dell'Europa e del mondo con inviti all'ONU ed al Parlamento europeo, il conferimento di premi, su tutti il "Templeton", per il progresso della religione ed il "Premio per l'educazione alla pace" nel 1986, oltre a molte, tantissime cittadinanze onorarie. Grazie all'impegno di Chiara Lubich oggi i focolarini sono diventati una grande realtà, presenti in 182 nazioni, con oltre 2 milioni di aderenti, con centocinquanta chiese cristiane e di varie religioni e città delle di testimonianza, sparse in tutto il mondo. La loro attività sociale si contraddistingue per importanti progetti, come ad esempio l'adozione, allo stato attuale, di ben 15.000 bambini a distanza. Un movimento diventato presto un popolo, una grande famiglia proprio come voleva Chiara Lubich, che oggi Maria Voce sta guidando con gli stessi princìpi che animavano la fondatrice. Colleghi senatori, ad un anno dalla sua scomparsa, invitiamo a guardare Chiara Lubich e le sue battaglie con gratitudine, ma anche con grande attenzione proprio per quanto oggi vediamo verificarsi davanti ai nostri occhi. Il dialogo tra le religioni è ancora una questione centrale per gli equilibri del mondo, spesso causa di conflitti e persecuzioni. Lei seppe anticipare i tempi, aprendo al confronto, superando steccati che sembravano insormontabili, affrontando platee diverse da quella abituali per conoscere, saper apprezzare, trovare punti di confronto anche nella diversità. Di fronte alla crisi economica ed al *crac* dei mercati finanziari, poi, le parole di Chiara Lubich, intrise di realismo e solidarietà non sono solo un monito, ma una concreta soluzione. Può esistere un modello diverso da quello consumistico e di sperpero imperante nella nostra società, che esclude gli ultimi, che mette al centro della vita il danaro ed il profitto e che si sta dimostrando in tutta la sua fragilità. Chiara Lubich ci ha indicato una via. Non limitiamoci a ricordare quanto ha costruito ma attualizziamo e facciamo fruttare i suoi inestimabili insegnamenti. Signor Presente, spero che ci sia silenzio anche solo per rispetto verso la figura di Chiara Lubich. Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, ricorre quest'anno, come lei ha detto, il primo anniversario della scomparsa di Chiara Lubich, fondatrice del Movimento cattolico dei focolari. Di Chiara, nel momento della conclusione del viaggio terreno ad 88 anni, in un clima sereno ma di intensa commozione, tra le parole più ricorrenti nella miriade di messaggi giunti da tutto il mondo, venivano indicate la luce e l'amore senza confini a testimonianza di una vita senza riserve. Tutto accade durante la Seconda guerra mondiale, a Trento, sotto i bombardamenti che fanno crollare ogni cosa. Chiara è lì, poco più che ventenne, ed in quel clima di odio e di violenza sperimenta l'incontro con Dio: il tutto, l'unico che per lei non crolla. Decide che vivere l'insegnamento puro e primigenio del Vangelo, accompagnandosi ai poveri dei quartieri più diseredati di Trento, seguendo l'esempio di Cristo, sarebbe stata la più potente rivoluzione sociale attuabile. Una scoperta da lei definita folgorante, più forte delle bombe che colpivano Trento, subito comunicata e condivisa dalle sue prime compagne. Nasce così il nucleo del movimento ecclesiale "Opera di Maria", meglio conosciuto come Movimento dei focolari, che per la varietà della sua composizione assume negli anni la forma di un popolo, di un vero laboratorio per un mondo unito nella fraternità. Si apre un nuovo orizzonte ed imprime una direzione decisiva, non solo nella vita di Chiara, ma in milioni di persone: l'intuizione che riscoprire il Vangelo avrebbe illuminato e rinnovato la società diviene lo scopo della vita di Chiara, interamente devoluta a concorrere e ad attuare il testamento di Gesù che tutti siano uno, il vero progetto di unità sulla famiglia umana. Negli innumerevoli volti del dolore, delle divisioni, dei traumi dell'umanità, Chiara riconosce il volto di Cristo, dell'uomo Dio che sulla croce grida l'abbandono del Padre: in lui trova la chiave per ricomporre l'unità tra Dio e gli uomini. L'unità tra singoli, categorie sociali e popoli, costantemente indicata come il primo impegno dell'intero movimento, è da lei alimentata con scritti, incontri e viaggi che richiamano sempre l'ispirazione e la radicalità originaria del carisma. L'incontro, come già detto, con il giornalista e deputato Igino Giordani, da Chiara ribattezzato "Foco" e ritenuto cofondatore del movimento per il suo contributo all'incarnazione nel sociale della spiritualità dell'unità, dimostra che l'esperienza del movimento è praticabile non solo da consacrati ma anche da sposati. Nelle fila dei focolari si possono annoverare uomini e donne delle più diverse categorie sociali, razze e culture: ai cattolici si uniscono cristiani di altre confessioni, ortodossi, anglicani, evangelico-luterani, ebrei, seguaci di altre religioni, buddisti, musulmani ed indù. Via via Chiara dà vita a modelli di una nuova socialità: le cittadelle che troviamo sparse nei cinque continenti, la prima a Loppiano Valdarno, presso Firenze. Per diffondere la cultura dell'unità moltiplica l'utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale. Il suo impegno per la creazione di nuovi modelli di socialità si rivolge ai più diversi ambiti della società. Nel 1991, di fronte agli enormi squilibri sociali del Brasile, dà vita al progetto delle economie di comunione; nel 1996 nasce il Movimento politico per l'unità, che propone ai politici delle più diverse estrazioni partitiche la fraternità quale categoria politica in vista del bene comune. Chiara si dedica ad aprire nuove prospettive per il dialogo ecumenico interreligioso e per la pace. È invitata a portare la sua esperienza in Thailandia, a New York, in Argentina. Ecco Chiara Lubich, questa figura femminile mite e forte che ha saputo illimpidire quel cielo grigio e cupo che ha attraversato l'intero Novecento. Una donna che ci interroga con l'attualità del suo messaggio, quasi fosse un'esortazione; una donna che ci invita a cogliere il senso del suo impegno, magari suscitando in noi una pretesa più alta, e perché no, facendoci sentire tutti un po' mendicanti di infinito. A me piace allora oggi immaginarla così, come quel germoglio che nell'approssimarsi della stagione che segue l'inverno riaccende la speranza, una ricchezza

colleghi, commemorare oggi Chiara Lubich per me è fonte di onore, ma anche di profonda commozione. Il suo messaggio nasce e si sviluppa da una fede profonda e senza riserve verso il Vangelo. La consapevolezza della propria fede e la sua universalità, le hanno fatto fare di Dio il perché della sua vita. Come aveva già citato anche lei, Presidente, Chiara negli negli anni Quaranta, all'età di vent'anni, prende atto che si viveva una situazione debolissima - c'era la guerra - e si rifugia nella fede: decide e capisce che bisogna fare qualcosa per questo mondo malato. Assieme a queste sue compagne decide di aiutare i poveri, facendo nascere il primo focolare, anche perché capisce che Dio gli dà la forza, l'illuminazione giusta per poter trasformare la sua esistenza e quella di tanti altri mostrandogli lo scopo di questa esistenza, che è concorrere ad attuare le

interamente immersa nella fede di Dio, nella consapevolezza anche di diventare e poi di essere uno strumento di Dio.

«Pur non essendo esperta in problemi economici, ho pensato che si potevano far nascere fra i nostri delle aziende, in modo da impegnare le capacità e le risorse di tutti per produrre insieme ricchezza a favore di chi si trova in necessità. La loro gestione è stata affidata a persone competenti, in grado di farle funzionare efficientemente e ricavarne degli utili, che lì sono veramente messi in comune.

«Ora tutto è veramente compiuto: il sogno degli inizi si è fatto verità, l'anelito appassionato è appagato: Chiara incontra Colui che ha amato senza vedere e piena di gioia può esclamare: sì, il mio redentore è vivo!».

Sicuramente auguro a Maria Voce, la persona che ha ereditato la gestione di questo grande movimento, una guida serena e

per questo bel momento; credo che il carisma di Chiara sia qui con noi e in mezzo a noi. Proprio lei diceva che anche i carismi migliori sono nulla senza la carità del cuore, una carità capace di appassionare l'anima, di illuminare la mente e di far definire il folle sogno di una ragazza che, a poco meno di 20 anni, comincia a vivere la sua vocazione e, com'è stato ricordato da molti e anche da lei, Presidente, da Silvia diventerà per sempre Chiara, Chiara Lubich, così come l'hanno conosciuta e amata anche molti di noi. Noi oggi la ricordiamo ad un anno della sua partenza - lei ha detto che raggiungeva il suo sposo - perché questa piccola grande donna ha segnato la storia del Novecento e ha impresso i suoi valori anche nelle aule del Parlamento; lo sta facendo oggi, ma l'ha fatto, con la dolcezza e l'autorevolezza che ha sempre contraddistinto Chiara, quando il 15 dicembre 2000 ha incontrato senatori e onorevoli a Palazzo San Macuto ed è stato lì - mi ed è stato lì - mi scuso per l'emozione - che ha lanciato questo grande movimento, un Movimento politico per l'unità, di cui fanno parte anche molti di noi. noi. È stata una ragazza come tante, cresciute nella povertà di un'Italia che stentava a riconoscersi, frastornata da guerre, povertà e malattie, che non dava spazio a vanità e e a volte nemmeno alla speranza, ma dove Chiara sperimenta la forza della fede, a Trento, sotto i bombardamenti, quando si ritrova con le sue prime compagne nei rifugi, leggendo il Vangelo e scoprendo le parole illuminate da una luce nuova. Per la prima volta fa breccia nel suo cuore il testamento di Gesù: «*Ut omnes unum sint*», che tutti siano uno, dal quale scaturisce proprio il carisma dell'unità. Quando i suoi genitori sono costretti a partire, lei decide invece di restare con le sue compagne, di stare in mezzo alla sofferenza. Proprio nella città natale nasce il primo focolare, qualcosa di intimo e familiare, capace di scaldare nel momento del bisogno e di radunare intorno ad esso la condivisione dell'amore e delle idee, il simbolo e la forza di un nuovo movimento, che ha avuto - è stato ricordato - anche l'approvazione del Papa. Come un piccolo seme, posto nel giardino della solidarietà e della fratellanza, con costanza e pazienza, Chiara ha annaffiato, giorno dopo giorno, ha resistito alle intemperie e ha gioito del sole, fino a veder nascere un albero le cui radici, forti e robuste, si sono diramate nel mondo, raggiungendo soprattutto i più deboli, i fragili e gli emarginati, ma è stata capace

la grandezza di Chiara era, ed è, proprio nella follia di quel sogno: portare a Dio il mondo fra le braccia, affinché tutti siano uno, Padre, come io e te. Chiara sapeva bene che le parole sono pietre, ma possono essere la vera forza dell'uomo per tradurre un abbraccio a distanza, per impedire le guerre, per far sorridere un bambino.

la fraternità riesce a declinare l'io nel tu e si eleva a categoria politica se, indipendentemente dalla provenienza, dalla religione e dall'appartenenza partitica, mira al bene comune. «La fraternità» - così diceva Chiara a Trento l'8 giugno 2001 - «se è necessaria dovunque, non può non esserlo nella politica. Perciò anche i politici, come tutti, sono chiamati ad impegnarsi a metterla in pratica ed a sentirsi fratelli fra loro, prima della stessa passione per il proprio partito, prima delle scelte che distinguono le diverse opzioni.

lasciando questo messaggio di Chiara: «Chiunque da solo si accinge oggi a spostare le montagne dell'indifferenza, se non dell'odio e della violenza, ha un compito immane. Ma ciò che è impossibile a milioni di uomini isolati e divisi, pare diventi possibile a gente che ha fatto della fraternità universale il movente essenziale della vita». La speranza di queste parole trova la loro finalità nel testamento di Chiara,

amatevi a vicenda, affinché tutti siano uno». Speriamo che questo amore sia presente anche tra di noi. Ribadisco Signor Presidente, desidero anche io ringraziarla non solo per il fervore che ha voluto riservare al ricordo di Chiara Lubich ma anche, come trentino, per aver voluto inserire in una mattinata così intensa di lavori

così quando Dio prende in mano una creatura per far sorgere nella Chiesa una sua opera, la persona non sa quello che dovrà fare». In questo momento, queste parole sono molto attuali e anche chi, in pochi minuti, deve ricordare lo straordinario percorso terreno di questa donna non sa quello che dovrà dire e nemmeno cosa dovrà scegliere nel formidabile e prezioso patrimonio di scritti che Chiara Lubich ha lasciato

Chiara Lubich è morta a 88 anni di età. In un mondo come quello attuale, che tutto brucia e consuma ogni giorno, la sua immagine e il suo carisma la rendono ancora vivissima nella sua sterminata famiglia che, come ricordato, è distribuita in tutto il mondo. Della sua biografia sono state già tracciate molte parti e molti passaggi ma vorrei ricordare come Chiara sia nata in una famiglia molto modesta. Il padre era un tipografo e sicuramente gli anni non erano dei migliori: infatti gli anni che precedevano il grande abisso del 1929 e, quindi, la vita era inevitabilmente molto modesta. Dalla madre, una fervente cristiana, ereditò la fede e dal padre socialista una viva sensibilità per tutte le vicende e gli aspetti della socialità. A 18 anni A 18 anni insegnava già tra i banchi delle elementari; poi si iscrisse all'Università, alla facoltà di filosofia a Venezia, ma la guerra, come abbiamo sentito dalle note biografiche già illustrate, la costrinse a lasciare gli studi. Abbiamo anche sentito come, proprio in un momento di grande difficoltà, sotto

Avrebbe poi detto nei suoi ricordi: «Quelle parole, prima quasi ignote, sono brillate come sole nella notte. Per quella pagina, noi siamo nate. Avevamo la certezza che Dio avrebbe trascinato la nostra vita in una divina avventura». Era davvero l'inizio di un'avventura che avrebbe raggiunto i confini del mondo e illuminato anche l'arte, la scienza, la politica e l'economia, attraverso una nuova corrente spirituale - la spiritualità dell'unità che rapidamente divenne universale, facendo leva sul principio che amore, unità e fraternità sono iscritti nel DNA di ogni uomo. Su questa spinta Chiara, come è stato già evidenziato, ebbe l'ispirazione di fondare il Movimento dei Focolari, che assunse rapidamente dimensione mondiale, coinvolgendo laici e sacerdoti, persone di ogni età, categoria sociale, razza e religione, catturate da nuove regole di vita: "uniti nella fraternità - che tutti siano uno - amatevi l'un l'altro come io ho amato voi". Poi, vi è stato un radicale salto di qualità «Perché l'umanità disgregata si ricomponga, mettiamo tutto in comune: cose, case, aiuti, denari, vita e destini, in una sola grande famiglia umana». Era solo il punto di partenza di un viaggio che avrebbe portato Chiara Lubich verso ulteriori orizzonti: quelli del dialogo ecumenico e del dialogo multireligioso.

In mezzo a persone non credenti e di varie ideologie, portò a casa - per così dire - come bottino di fede ben 70.000 persone che aderirono al Movimento, là dove non vi erano - ripeto - né fede né credenze. Il dialogo poi si estese alla cultura: sin dagli inizi del Movimento, Chiara aveva intuito che il carisma dell'unità avrebbe avuto un impatto anche in questo mondo. Nacque così la Scuola Abbà, forte del carisma dell'unità, dove docenti universitari ed esperti di varie discipline si impegnarono ad elaborare le prime linee di una cultura nuova, più illuminata.

Intanto, nella cittadella di Loppiano, che è stata ricordata, nasceva l'Istituto universitario Sophia, inaugurato l'anno scorso. Voglio ricordare anche il suo viaggio in Brasile: colpita dagli enormi squilibri economici e sociali di quel Paese, diede il via al progetto dell'economia di comunione, che ancora oggi ispira la gestione di oltre 700 aziende di produzione di beni e servizi, che destinano parte dei loro utili ai meno abbienti. Infine, l'ultima annotazione, non secondaria, riguarda la nascita del Movimento politico per l'unità, nel 1996, al quale aderiscono oggi soggetti politici delle più diverse estrazioni, in molti Paesi del mondo, accomunati dalla fraternità assunta come categoria politica. Al nostro momento commemorativo, fino a pochi minuti fa, assistevano

da sentimenti di fraternità, pur divisi da differenze di carattere politico. Ma sui valori fondamentali proprio il valore dell'unità prevale su qualsiasi differenziazione. Ieri e lunedì alla Camera, oggi qui al Senato la testimonianza anche di questi parlamentari, venuti appositamente in occasione del primo anniversario della morte di Chiara Lubich da ogni angolo del mondo, costituisce un contributo straordinario al ricordo di Chiara Lubich e sono essi la garanzia vivente il suo messaggio di unità universale non avrà cedimenti, così come il suo patto di fraternità per l'Italia, che la collega Emanuela Baio ha ricordato poco fa, consegnato ai parlamentari italiani a San Macuto nel 2000, recitava: «Un patto che metta il suo bene» - il bene dell'Italia - «al di sopra di ogni interesse parziale, sia esso individuale, di gruppo, di classe o di partito». insomma, una visione alta della politica, destinata a mantenere vivo ed attuale il carisma di Chiara Lubich per molto, molto tempo ancora, forse per sempre. Si conclude così questo significativo momento commemorativo che il Senato ha voluto dedicare a Chiara Lubich, ad un anno dalla sua scomparsa.

per cento dei voti ottenuti. Questo perché la modifica alla legge elettorale europea aveva implicitamente, e non esplicitamente, innalzato questa soglia al quattro

soffermerò in sede di replica, se sarà necessario. Tuttavia, l'articolo 5 del decreto prevede una copertura di 1.451.850 euro, non perché il saldo del provvedimento, una volta applicato, sia negativo, ma perché le spese aggiuntive sono determinate dagli adempimenti per agevolare il voto dei nostri connazionali temporaneamente all'estero, mentre non può essere conteggiato il risparmio che viene ottenuto dall'accorpamento

le elezioni amministrative al 6 ed al 7 giugno, in coincidenza con le elezioni europee.

Nell'ansia di motivare la richiesta con un possibile risparmio per le casse dello Stato, avevano omesso di dire che in quel caso

deputati. Onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento - il quale prevede che il Senato discute e delibera soltanto sulle modificazioni apportate apportate dalla Camera dei deputati - comunico che sono inammissibili l'ordine del giorno G1.1 e gli emendamenti 1.1 e 1.0.2, in quanto non fanno riferimento né si trovano in correlazione con l'unica modifica introdotta dalla Camera dei deputati, dei deputati, relativa alla soppressione dell'articolo 1-*bis* sui contributi per le elezioni europee. Presidente, so bene che la decisione della Presidenza sull'inammissibilità dell'ordine del giorno è inappellabile, però mi permetta di svolgere alcune considerazioni di segno assolutamente contrario rispetto a tale pronuncia di inammissibilità.

all'attività di emenda del testo e quindi non è un criterio per valutare l'ammissibilità - o l'improponibilità, forse, *rectius* - di un ordine del giorno. L'ordine del giorno, secondo l'articolo 97 del Regolamento, per essere ammissibile non deve essere estraneo all'oggetto della discussione, né formulato in termini sconvenienti. Un ordine del giorno con il quale si impegna il Governo ad accorpare alle elezioni amministrative ed europee anche le consultazioni referendarie per evitare di buttare dalla finestra circa 400 milioni di euro

anche perché quelle previste dall'articolo 97 sono prescrizioni di restrizioni che riguardano il diritto del parlamentare ad intervenire su provvedimenti in discussione e quindi non possiamo dare loro né un'interpretazione analogica, né tanto meno un'interpretazione estensiva. Peraltro stiamo discutendo di un disegno di legge di conversione di un decreto-legge, quindi ci esprimiamo su un articolo unico. Ovviamente nelle dichiarazioni di voto e nella discussione generale non c'è un limite, se vogliamo ancora prendere a riferimento l'articolo 104, a che la discussione verta su parti del provvedimento che non sono state modificate. Tra l'altro si tratta di un ordine del giorno riferito al contenuto generale del provvedimento e quindi la preclusione dell'articolo 104 del Regolamento non può estendersi in via analogica alla presentazione di un ordine del giorno dello stesso

bilancio il Governo si è di fatto rifiutato di fornire una quantificazione del risparmio che deriverebbe dall'accorpamento della consultazione referendaria con le consultazioni amministrative e le elezioni e le elezioni del Parlamento europeo. Siccome non c'è una spiegazione in ordine a questo fatto e siccome l'ordine del giorno verte sul risparmio di una somma considerevole che può essere utilizzata ben altrimenti che per la fissazione di una data ulteriore per lo svolgimento del *referendum*, francamente ritengo che la decisione della Presidenza di considerare inammissibile l'ordine del giorno G1.1, mentre è perfettamente coerente con i silenzi imbarazzati del Governo in ordine ad una domanda da noi esplicitamente posta in Commissione bilancio, sia incompatibile con l'applicazione degli articoli 97 e 104 del Regolamento.

«se un disegno di legge approvato dal Senato è emendato dalla Camera dei deputati», come nel caso in questione, «il Senato discute e delibera» - non delibera soltanto, quindi - «soltanto sulle modificazioni apportate dalla Camera». In senso proprio, pertanto, le materie che non sono state modificate nella navetta tra Senato e Camera sono estranee all'oggetto di discussione e, in relazione ad esse, non è consentita la presentazione di strumenti che conducono ad una votazione (emendamenti o ordini del giorno), poiché non si può votare ciò che non è possibile discutere. Questa è stata l'interpretazione che ha assunto la Presidenza. Tuttavia, come si è visto, la Presidenza, nel consueto spirito di collaborazione con i colleghi senatori, ha dato la parola alla presidente Finocchiaro, che ha fatto riferimento all'ordine del giorno, pur non potendo avendo deciso la non ammissione di quest'ultimo alla votazione.

Presidente, l'emendamento 1.0.1 evoca, in verità, il testo approvato dal Senato nella prima lettura che alla Camera dei deputati è stato invece

che ha parzialmente ricordato quel passaggio - aveva invece sottolineato e cioè la necessità di differenziare le due soglie: quella per

prima riguarda la spesa: vi è stata qualche polemica, anche su importanti organi di stampa, sull'eventualità che quell'emendamento, che a suo tempo passò al Senato e che poi la Camera respinse,

per accedere ai rimborsi elettorali basta lo 0,5 per cento, perché i due temi (la rappresentanza istituzionale e la rappresentanza politica), come sanno non solo i politologi, ma tutti i colleghi e le colleghe, sono colleghi e le colleghe, sono concetti contigui ma diversi. Si può avere una forza politica senza rappresentanza istituzionale

un aspetto che è stato suscitato dalla presidente Finocchiaro sulla questione del costo del non accorpamento del turno referendario con le elezioni amministrative. Su questo punto, anch'io avrei la curiosità di sapere quale sia la stima da parte del Governo e mi permetto di sottoporne una basata sulle uniche cifre che si possono conoscere: il compenso che avrebbero

di 97 euro per il presidente e di 82 euro per ciascuno degli scrutatori. Avremo quindi un totale

gli straordinari dei dipendenti comunali ed altre spese, arrivando così, a mio modesto parere, ad un totale di circa 40 milioni di euro. Se non è così, credo sia bene saperlo, perché vuol dire che forse c'è qualche diseconomia nella gestione della procedura elettorale. Ma credo che la cifra di cui stiamo parlando sia di 40 milioni di euro, che è stata generosamente, ma so diffusamente, invece, stimata in 400 milioni

Il *referendum,* le elezioni amministrative e quelle politiche hanno costi differenti, in parte a totale carico dello Stato, in parte a carico delle amministrazioni locali. In parte si tratta

perché sapevo di compiere un gesto velleitario in quanto quello che di politicamente sostanziale era avvenuto sappiamo coglierlo. percepito una disponibilità, che si era tradotta nell'accoglimento della proposta in Senato; abbiamo preso atto di una revisione profonda

la norma relativa al rimborso elettorale. È stato particolarmente utile l'intervento del collega Vita perché ha distinto, in modo molto chiaro, il tema della selezione della rappresentanza dalla questione della competizione democratica alle elezioni. Il rimborso elettorale è uno strumento essenziale per la vita democratica e per la gestione trasparente dei partiti, soprattutto di quelli piccoli che non hanno la possibilità di accedere a forme di finanziamento importanti o perché non godono di soci sostenitori corposi nella loro forza finanziaria o perché non godono dell'attenzione di grandi gruppi economici che dell'amicizia

fondata tutta sul rimborso elettorale. Una trasmissione televisiva ha pure reso noto che la Lega Nord ci riversa una quota di finanziamento di 293.000 euro come se fosse un atto scandaloso. in modo chiaro e trasparente la quota di finanziamento relativa alle elezioni del 2006 in cui, alleati con la Lega Nord, per la parte di consenso che abbiamo contribuito ad ottenere nel nostro territorio, facendo di conto, secondo regole chiare ed aritmetiche, abbiamo avuto titolo per quel finanziamento. Quindi non era né una graziosa concezione né un atto clandestino, ma un atto chiaro, politico, trasparente su cui si fondava l'intesa elettorale tra noi e la Lega Nord.

di attenzione relazionale con le forze più piccole della coalizione perché la soglia di sbarramento al 4 per cento, come ha spiegato bene il relatore, ha determinato un innalzamento drastico per l'accesso al finanziamento, per una campagna elettorale, quella per le europee, impegnativa dal punto di vista della comunicazione e quindi anche molto, molto onerosa.

per recuperare risorse a carico del pubblico erario. Era una quota politica cui potevano avere accesso soltanto forze organizzate o per esperienze territoriali o culturali già sufficientemente rilevanti. La scelta drastica compiuta alla Camera conferma questo processo di semplificazione. Dico una battuta: di semplificazione in semplificazione, la democrazia si restringe ed assumo serenamente la responsabilità di questo argomento perché impedire condizioni di partecipazione democratica in una campagna elettorale è una scelta miope. Essere partiti di maggioranza comporta un di più di responsabilità.

ma deve consentire la partecipazione e la competizione, garantendo l'accesso alla rappresentanza. Dopodiché, è giusto che le regole di filtro per la rappresentanza parlamentare a sostegno del Governo siano legate siano legate a princìpi di efficienza. Ma è stato un grandissimo errore. Io credo, caro relatore, che la sua riflessione imbarazzata, il voler ricondurre la sua la sua scelta ad un principio di acquiescenza a quello che è stato deciso alla Camera di deputati sia anche un limite ed un errore istituzionale. Troppe volte il Senato subisce la primazia politica della Camera dei deputati. Capisco che forse per voi non è questo il caso in cui far valere il

forse, vi è la capacità di un di più di riflessione quantomeno per ragioni numeriche. Siamo di meno e ragioniamo di più. Almeno spero che sia così. Per questo dichiaro il mio voto favorevole all'emendamento 1.0.1, preannunzio anche il voto contrario al complesso del provvedimento.

È pervenuta alla Presidenza una riformulazione dell'ordine del giorno G1.1, presentato dalla senatrice Finocchiaro e da altri

alle modifiche che sono state introdotte dalla Camera. Potrei dire semplicemente - ho consultato il presidente Schifani ed egli è d'accordo - che questo elemento di valutazione, per chiarezza con l'Aula, è come se non ci fosse. In coscienza, al di là del fine o delle convinzioni politiche, che sono altra cosa,

*(PD)*. Signor Presidente, credo che la sua decisione sia tecnicamente sbagliata. Lei aveva certamente ragione - ed ha avuto ragione la Presidenza del Senato - quando ha dichiarato inammissibile l'ordine del giorno nella sua precedente formulazione, poiché risultava evidente che esso non

è evidente che tra le ragioni che hanno indotto la Camera dei deputati a modificare il testo approvato dal Senato, ne può essere individuata una relativa all'introduzione di un risparmio. È del tutto evidente, infatti, che la norma approvata dal Senato, a proposito di finanziamento delle campagne elettorali, aveva un carattere che allargava la platea degli aventi diritto al finanziamento, rispetto al testo che adesso la Camera ci viene proponendo. Senatore Malan, soltanto un pregiudizio può indurla a sostenere il contrario. È chiaro che, con la modificazione apportata dal Senato, la platea dei beneficiari era più ampia, mentre è del tutto evidente che a questo punto, dopo la modificazione della Camera, la platea dei beneficiari è più ristretta. Poiché l'introduzione di un risparmio, rispetto al testo introdotto dal Senato,

Al primo passaggio di questo decreto al Senato, la delegazione radicale (parlo quindi anche a nome della senatrice Poretti) si è astenuta, perché alcune delle nostre preoccupazioni sono state

qualificherà per la storia della letteratura politica del nostro Paese questo decreto relativo al cosiddetto *election day.* Non ultima è la questione dei soldi: non si è riusciti neanche a mettere nero su bianco la necessità di documentare le spese relative alla campagna elettorale. Il senatore Pistorio ha giustamente parlato poco fa di finanziamento pubblico dei partiti, mentre invece la legge prevede un rimborso elettorale. Sarebbe utile, visto e considerato che in molti, anche qui dentro, continuano quotidianamente a stracciarsi le vesti relativamente alla necessità di essere trasparenti o di essere l'unica opposizione nei confronti di questa maggioranza,